sono stati apportati tagli pesanti al settore dell'università, della ricerca e della scuola. Faccio soltanto una rapidissima esemplificazione. il fondo di finanziamento ordinario dell'università, che è il fondo che regola la vita delle università. Vengono tagliati i fondi per la programmazione e la valutazione della politica universitaria e della ricerca. Vengono tagliati i fondi per i piani triennali di sviluppo dell'università, per l'edilizia universitaria, per il diritto allo studio, per le residenze e gli alloggi degli studenti. Vengono tagliate risorse per la ricerca e anche persino per la scuola.

anche che dopo l'infausto provvedimento Mussi, il regolamento sul reclutamento dei ricercatori che ho già ho avuto occasione di denunciare e che se dovesse entrare in vigore farebbe sì che

L'emendamento, fra l'altro, è stato presentato dal relatore, il senatore Benvenuto. Devo dire, senatore Benvenuto, che lei un tempo fu vicino a Craxi, ma egli ebbe ben altra attenzione verso l'università. Voi state tradendo tutte

se fosse un fatto squisitamente veneto, un banale litigio tra Veneto e Trentino-Alto Adige. Presidente, non è così, la questione è molto più grave e occorre che venga il Governo a riferire in Aula. Aula. Fino ad oggi il Governo è rimasto a guardare, mentre si cerca di ridisegnare la geografia del Nord Italia in base a questioni di carattere prettamente economico... PRESIDENTE. Senatrice, possiamo parlarne in chiusura di seduta. Cortina appartiene al Veneto e l'invito alla secessione fatto dal governatore altoatesino Durnwalder è un atto eversivo, oltre che insopportabile. Chiediamo quindi la presenza del Governo

*(LNP)*. Signor Presidente, onorevoli colleghi, la Conferenza internazionale sullo stabilimento dello Stato di diritto in Afghanistan, che si terrà a Roma il prossimo 3 luglio, scuote la sensibilità del Senato: è un fatto altamente positivo che siano stati prodotti per l'esame in quest'Aula quattro mozioni e più ordini del giorno. Il nostro Paese - lo sappiamo l'impegno particolare della riforma della giustizia e, fino al gennaio 2006, l'Italia è stata *lead* *country*, mentre oggi ricopre il ruolo di coordinatore di questo settore,

afghana (che oserei definire quasi impossibile nella sua attuazione). Esporrò, a beneficio dei colleghi tutti, le mozioni presentate dal mio Gruppo, facendo ricorso e riferimento alle nozioni e notizie apprese attraverso la Commissione esteri, di cui faccio parte. *(Brusìo).*

Economist», per il suo ultimo dettagliato servizio dall'Afghanistan - lo dico soprattutto a beneficio del senatore Salvi

È una definizione che ben inquadra le serie difficoltà incontrate sul terreno del programma di riforma intrapresa più di quattro anni fa dal nostro Paese. Lega Nord è ben consapevole che, ancor più che una condizione di difficoltà, ciò che è da superare e vincere è la precisa circostanza che in quel Paese asiatico, grande quanto l'Italia e la Francia, è l'assenza di una struttura radicata a livello locale, in grado di contrapporsi dialetticamente allo strapotere del codice tribale che rende impossibili i tentativi della comunità internazionale di affermare la *rule* *of* Ulteriore difficoltà oggettiva, signori colleghi, colleghi, è data dal fatto che la Costituzione afghana, approvata nel 2004, fa riferimento sia alla legge civile sia alla *sharia* islamica: questo punto di partenza non può essere né sottovalutato né tanto meno dimenticato. Dopo anni di profusione d'impegno, la situazione del programma giustizia si può dire, signor Presidente del Senato, essere ferma al palo e quella vale a dire che ci rappresenta al «The Economist» attraverso il suo dettagliato servizio. E io dico, per quel poco che mi è stato dato di apprendere e capire, che non può e non poteva essere diversamente, ove si tenga conto che in Afghanistan, paese musulmano e dalle forti tradizioni, vigono, signori senatori, tre differenti sistemi giuridici, cioè sono in atto, sono operativi, regolano la vita del Paese e dello Stato, tre differenti sistemi giuridici: il diritto civile (in parte simile a quello della Turchia, dell'Italia e della Svizzera), la legge islamica e il diritto consuetudinario o «materiale». Rispetto a tale triplicità di sistema giuridico occorre essere consapevoli, signor Presidente del Senato, che il «diritto materiale» è tuttora basato sui codici tribali che prevalgono su qualsiasi tentativo di formalizzazione ed applicazione della *rule of law*. Tali codici tribali, signori della maggioranza soprattutto così ansiosi di non voler sentire,

si autolegittimano come propriamente islamici grazie al riconoscimento loro fornito a suo tempo dal regime dei talebani, in contropartita delle alleanze territoriali strette con tribù, allora, delle varie etnie. Di modo che, ed ecco la conclusione dello stato delle cose, è possibile ripetere oggi ciò che sostengono osservatori bene addottrinati ed attenti: dopo cinque anni dalla caduta del regime talebano la maggior parte delle incriminazioni e sentenze che portano alla detenzione risponde ancora, sostanzialmente, alla logica dei codici tribali, ripeto, egregio senatore Salvi - mi spiace doverglielo dire io che non sono giurista come lei - risponde sostanzialmente alla logica dei codici tribali. Poi c'è un'altra questione che

un popolo dalle tradizioni plurisecolari può approdare alla modernità?» Con lealtà è forse il caso di chiederci se i valori di democrazia dei diritti umani non vadano presentati e rappresentati al popolo africano in modo da renderli almeno moderatamente coniugabili con quelli arcaici e tradizionali degli africani medesimi, da noi ritenuti inaccettabili a ben ragione, dal nostro punto di vista. Ma penso e con me ne è convinto il mio Gruppo parlamentare - che si proceda da parte nostra in spirito di grande comprensione e, ancor più, di grande tolleranza verso quella popolazione e le autorità afgane. Prova evidente di ciò è riscontrabile nell'acquiescenza del nostro Paese rispetto alla decisione delle autorità africane per quanto concerne il codice di procedura penale, di averlo rinnovato, in quel Paese, ed approvato *ad interim*, ovvero provvisoriamente, e con scarsa possibilità di apporto oltre che nostra di italiani anche del resto della comunità internazionale; di avere noi tollerato, noi che siamo lì in funzione di uno stabilimento di quadro giuridico e giudiziario nuovi, che quel Paese approvasse gli stessi identici contenuti e articolati vigenti antecedentemente al regime talebano, rifiutando ogni altra (nostra e della comunità internazionale) indicazione. Di fronte a tale kafkiana situazione, il Gruppo cui appartengo con le sue mozioni si è posto sul piano di massimo realismo, ben consapevole che se per un verso l'impegno riformatore della giustizia afghana è irto di difficoltà, per altro verso è un impegno che deve produrre effetti positivi. Direi con sensibilità umana, con intelligenza politica, con senso di opportunità strategica il mio Gruppo, attraverso le sue mozioni, muove precise sollecitazioni. luogo, impegna il Governo italiano a cogliere l'occasione della prossima Conferenza internazionale di Roma per reimpostare una nuova fase della *rule of law* in Afghanistan, stringendo, per una più efficace e sentita partecipazione ai lavori, le autorità afgane e l'intera comunità internazionale interessate. Impegna, per altro verso, il Governo italiano ad opporsi alla partecipazione a future Conferenze internazionali di Paesi fornitori di armi a sostegno ai movimenti terroristici internazionali. inoltre il Governo italiano a riconsiderare in radice il problema della gestione dei sequestri di persona, in particolare chiedendo che il Governo non negozi più riscatti o scambi di prigionieri nel corso di rapimenti di cittadini italiani all'estero. Per

Mi preme fare una qualche considerazione molto veloce, e non perché voglia portare critica a ciò che altri Gruppi, altri presentatori di mozioni, pienamente, autonomamente e legittimamente

dell'osservanza della discrezione e del rispetto del prossimo, però mi pare che questa mozione veramente ce la metta tutta per per fare uscire da uno schema di rigore metodologico di un approccio sereno e riguardoso verso gli altri e far dire: che cosa si vuole intendere in tutta questa enorme premessa di una mozione, che poi si compendia in tre postulati, in tre postulati, che si scopre ancora l'acqua fresca? Scusatemi, dico questo non perché voglia mancare di riguardo, ma perché per economia di tempi devo anche rendere l'idea di ciò che voglio dire. Si pone alla prossima Conferenza di Roma la necessità che si veda come urgenza l'attuazione di una profonda riforma che possa contribuire a creare un clima di certezza di diritto. Ma allora non si conosce la situazione afghana dal punto di vista regolamentare, del diritto, della normativa, che è tale da far dire ad un osservatore attento come l'ambasciatore Vendrell che lì vige una situazione per cui, già al di fuori dello stretto perimetro della città di Kabul lo Stato non esiste, lo Stato è completamente assente, inesistente. Quindi, si usa una terminologia come se si trattasse di un Paese munito di un quadro giuridico sufficientemente certo e di cui si reclama maggiore certezza del diritto: ma questo è veramente fare demagogia gratuita. Si impegna il Governo ad un ad un programma di riforma della giustizia, accompagnato da un programma altrettanto robusto per la tutela ed il ripristino dei diritti umani: non sono conseguenziali, non è uno il postulato e l'altro il corollario, non è il quadro giuridico premessa indispensabile, la condizione *sine qua non* per un quadro di rispetto dei diritti umani e civili? Ma, allora, di che cosa stiamo parlando? Ma, allora, per quale motivo si è indetta la Conferenza internazionale di Roma del 3 luglio? del 3 luglio? Non pensiate di strumentalizzare anche istituti e istituzioni così importanti,

di una Comunità internazionale per questi Paesi. Non pensiate di fare della Conferenza di Roma un qualcosa che ponga al centro le questioni di Gino Strada, dei suoi amici e dei suoi compagni,

non pensiate di poterlo fare attraverso questi strumenti, sono finiti i tempi del Sessantotto, siamo ormai su un altro pianeta e in un'altra era. signor Presidente, grazie della pazienza, vado a concludere. Sono anch'io per la riconciliazione nazionale. D'altra parte, le mozioni della Lega vanno in questo senso. Ripeto, per ognuno che abbia comune buonsenso, il presupposto della riconciliazione nazionale sta in un quadro giuridico di certezze e noi siamo per questo. Però attenzione a questa smania di trotzkista memoria delle commissioni d'inchiesta, dal medioevo in poi quasi, attraverso le quali poi far seguire le pene severe; mi sa tanto di tempi passati, mi sa tanto di tribunali speciali.

Sottolineo che, da intese prese nella riunione dei Capigruppo, stiamo facendo una discussione che ingloba anche le dichiarazioni di voto. È iscritto a parlare il senatore Barbato. Ne ha facoltà. Signor Presidente, colleghi, la Conferenza sulla giustizia in Afghanistan, indetta a Roma per il prossimo 3 luglio, rappresenta un appuntamento di altissimo profilo da intendere, come qualcuno in questi giorni ha scritto, quale possibile «battesimo dell'Afghanistan come Stato di diritto, non solo più fragile alchimia istituzionale». L'Italia riveste il ruolo di relatore nella Conferenza per il delicato compito affidatole, sulla base dell'Accordo di Bonn del 2001 e delle successive conferenze che hanno delineato il percorso per la ricostruzione delle istituzioni statuali dell'Afghanistan, di guida per la ricostruzione del sistema giudiziario nel Paese, insieme alle autorità afgane e all'UNAMA (ente dell'ONU preposto alla ricostruzione del Paese). [**Presidenza *lead country* (Paese guida) per l'assistenza al Governo afghano nell'opera di ripristino di uno Stato di diritto, condizione essenziale per la nascita di una democrazia e, in particolare,

nel Paese nel rispetto degli *standard* internazionali dei diritti umani. Il nostro Paese ha, dunque, il delicato compito di fornire un'assistenza tecnica qualificata al Governo di Kabul, nel rispetto della sua sovranità. Al contempo, ha il dovere di esprimere una posizione forte e chiara circa la necessità che le autorità afgane osservino il pieno rispetto dei diritti umani e dei trattati internazionali ed il superamento definitivo di processi che, pare, in alcuni casi continuino a svolgersi secondo il codice tribale. Le autorità afgane devono sicuramente tentare la complessa (ma certo non impossibile) conciliazione delle sue tradizioni, della *sharia*, con il rispetto dei trattati internazionali. Alcune strade si stanno già utilmente percorrendo: penso, ad esempio, alla redazione del codice di procedura penale, del codice minorile e delle leggi penitenziarie, grazie al contributo fondamentale prestato dall'Italia. Molti altri obiettivi ancora, però, restano da perseguire. Mi riferisco, in particolare, alla fondamentale riabilitazione delle istituzioni della giustizia, cioè del Ministero della giustizia, della Corte suprema e della procura generale, la formazione di giudici, procuratori, avvocati e quadri direttivi del Ministero della giustizia. Un ultimo accenno al caso di Rahmatullah Hanefi: vorrei esprimere, anzitutto, soddisfazione per l'esito della vicenda e il riconoscimento dell'efficace azione diplomatica condotta dal Governo italiano. Il caso Hanefi è emblematico del fatto che, laddove non sussista un clima di certezza del diritto, possa essere incriminato chiunque sulla base di qualche sommario indizio, quindi senza una concreta imputazione, e recluso in condizioni di detenzione ignote. Ci auguriamo davvero - ed il Governo italiano dovrà spingere in questa direzione - che in Afghanistan venga segnata una seria svolta per quanto riguarda anche la situazione delle carceri e che sia riservata una particolare attenzione alle condizioni di giovani donne e bambini che vivono in condizioni drammatiche istituendo percorsi di riabilitazione e programmi di assistenza. PRESIDENTE.

condividendo la preoccupazione diffusa in tutto il Paese per la difficile situazione dell'Afghanistan. A distanza ormai di sei anni dall'intervento armato che ha rovesciato il regime dei talebani e ha avviato un difficile contrasto con il terrorismo qaedista, dopo la tragedia dell'11 settembre 2001, la situazione nel la situazione nel Paese afghano è tutt'altro che pacificata e risolta. In particolare, abbiamo espresso grandissima preoccupazione per gli episodi di scontro che hanno visto coinvolte anche le nostre Forze armate nell'area assegnata al nostro contingente, e quindi nord-occidentale del Paese, di poche settimane fa. Sono stati episodi molto gravi perché hanno evidenziato tutta la debolezza della strategia di contrasto al terrorismo che si sta conducendo in quel Paese. Per lungo tempo l'Afghanistan è stato diviso in due zone: quella del lungo confine con il Pakistan, dove si concentravano gli scontri armati,

Gli scontri che si sono svolti nella zona di Herat, dove si trova il nostro contingente, hanno invece infranto questa fragile convinzione ed hanno evidenziato il rischio che la guerra dilaghi in tutto il Paese e renda molto difficile il perseguimento di un'azione di *peacekeeping*. Infatti, è del tutto evidente che si tratta di una guerra, in particolare condotta con l'arma aerea, che fa molta fatica a discriminare e a distinguere tra forze terroristiche o forze comunque ostili al Governo Karzai e popolazione civile. Si tratta di uno strumento del tutto inadeguato a contrastare in maniera efficace la presenza e l'infiltrazione di forze estremiste, fondamentaliste e insorgenti; anzi corre il rischio veramente grave di provocare una saldatura tra la popolazione civile, che continua a soffrire di vittime innocenti e spesso indiscriminate di bombardamenti aerei in modo particolare, e le forze terroriste.

è quella di un negoziato internazionale. Abbiamo parlato più volte, anche in quest'Aula, di Conferenza internazionale sull'Afghanistan, una Conferenza che naturalmente deve vedere protagonista innanzi tutto il Governo Karzai.

su cui si gioca la prospettiva di costruire in Afghanistan uno Stato degno di questo nome e dunque un sistema istituzionale che possa dare gambe e scheletro alla fragile, oggi fragilissima, democrazia afghana. Credo pertanto che non si possa non guardare con soddisfazione e con simpatia a questa importante iniziativa internazionale che ha visto e vede il nostro Governo in una posizione di assoluto protagonismo.

ad una più ampia serie di colloqui a livello internazionale per una uscita ragionevole dalla crisi afghana. L'urgenza e la necessità di una riforma del sistema di polizia e di quello giudiziario in Afghanistan sono state rese ulteriormente evidenti dalle vicende che hanno coinvolto Emergency e in particolare il mediatore che fu impegnato nella difficile ricerca di una soluzione umanitaria al rapimento del nostro concittadino, il giornalista de «la Repubblica» Daniele Mastrogiacomo, del suo autista e del suo interprete. Sappiamo che Mastrogiacomo è stato felicemente restituito al nostro Paese, alla sua famiglia, al suo lavoro; sappiamo altrettanto che purtroppo questo non è avvenuto per gli altri sequestrati e sappiamo anche che c'è stato uno strascico, una coda di sofferenza che ha riguardato proprio il mediatore di Emergency che si era attivato in modo particolare per la felice soluzione di questa vicenda.

Non si tratta soltanto di una ragione umanitaria o di una ragione di solidarietà con una persona che comunque si era spesa a favore di un cittadino italiano: si tratta di difendere una delle ragioni fondamentali per le quali siamo lì. Sarebbe ben strano se noi fossimo in una lotta contro il terrorismo islamista e fondamentalista che conduciamo proprio in ragione dei diritti umani e poi vedessimo negare questi stessi diritti umani da parte del Governo e delle autorità che abbiamo sostenuto e che continuiamo a sostenere convintamente. Il positivo esito della vicenda naturalmente è per noi motivo di grande soddisfazione, ma il suo protrarsi nel tempo ci ha rafforzato nell'idea che è necessario esercitare la massima pressione perché perché l'Afghanistan possa vedersi finalmente riconosciuto un sistema giudiziario degno di quella Dichiarazione universale dei diritti dell'uomo

il presidente della Commissione giustizia senatore Cesare Salvi. L'impegno quinquennale assunto dall'Italia nel sostenere la riforma del sistema giudiziario in Afghanistan, impegno che prevede, come è noto, lo stanziamento di risorse pari a circa 50 milioni di euro, è uno dei punti qualificanti del piano di cooperazione e sviluppo che vede coinvolto il Governo italiano insieme ad altri. Va detto subito che tale impegno era per molti versi obbligato, considerata la situazione di estremo degrado in cui versa il settore della giustizia in Afghanistan, e dettato dall'urgenza di creare un clima di certezza del diritto nel Paese, condizione essenziale, quest'ultima, per ipotizzare un'effettiva pacificazione e riconciliazione nazionale. Tuttavia, sarebbe scorretto ignorare come si sia fin qui registrato un sostanziale fallimento di tale progetto, vanificato prima dal lassismo delle istituzioni afghane che poco o nulla hanno fatto per darne attuazione, tant'è che esso giace tuttora nelle commissioni miste di esperti afghani e internazionali - e poi ridicolizzato dalla vicenda che ha coinvolto il funzionario dell'organizzazione umanitaria Emergency, Rahmatullah Hanefi, vicenda i cui tormentati sviluppi hanno dimostrato quanta strada vada ancora percorsa sul piano del rispetto e della tutela dei diritti umani fondamentali. In effetti, la detenzione illegale di Hanefi, il quale per conto del Governo italiano ha svolto un ruolo decisivo di mediazione per la liberazione del giornalista de «la Repubblica» Daniele Mastrogiacomo e, prima ancora, del *freelance* Gabriele Torsello e, nonostante ciò, incriminato con le farneticanti accuse di «contiguità con Al Qaeda» formulate dal Governo Karzai, pesa come un macigno sulle prospettive future della giustizia afghana. È impossibile dimenticare che quest'uomo ha trascorso tre mesi in totale isolamento, in un luogo sconosciuto, senza poter incontrare un avvocato e senza che fossero rese note le accuse a suo carico né gli indizi che hanno portato alla sua incriminazione. Così come è impossibile sottacere che tale episodio ha messo a grave rischio la sicurezza di tutto il personale di Emergency, obbligando l'ONG a rinunciare all'impegno che da nove anni svolgeva in Afghanistan, assistendo oltre un milione e mezzo di persone, prevalentemente bambini e civili. E, paradossalmente, il fatto che egli sia stato infine scarcerato, grazie soprattutto alla fortissima pressione esercitata dalla società civile internazionale, senza che a suo carico sia stato reperito il benché minimo elemento di colpevolezza, aggrava ulteriormente la condotta del Governo Karzai che - è bene ricordarlo - ha ripetutamente sostenuto che la detenzione di Hanefi era un atto dovuto in considerazione degli indizi raccolti a suo carico. Che cosa sarebbe successo, viene lecito chiedersi, se non si fosse verificata una mobilitazione così massiccia per ottenere la sua liberazione? Non è azzardato ritenere che, nonostante la sua assoluta innocenza, Hanefi sarebbe potuto rimanere segregato a tempo indeterminato nelle carceri afghane se non, addirittura, essere giustiziato, come più volte minacciato da fonti, non si sa quanto attendibili, di Kabul. Dunque, su questa vicenda penso sarebbe opportuno tornare in occasione della Conferenza internazionale di Roma del 3 luglio: quel che è accaduto è, infatti, indice di una cultura del diritto ancora allo stato embrionale, di cui è opportuno mettere in evidenza tutti i limiti anche per garantire che organizzazioni come Emergency possano in futuro svolgere in piena tranquillità e sicurezza il proprio lavoro, perché se è vero che è importante il tema giustizia, è altrettanto vero che in quel Paese in particolare è centrale il tema della salute e della sanità. Ma molti altri punti dovrebbero essere dibattuti alla Conferenza, come quello concernente, ad esempio, la grave situazione, confermata anche da recenti rapporti sul campo, riguardante il penitenziario di Pol-i-Chark, finanziato dal Governo italiano e situato a 25 chilometri da Kabul. Questa struttura è attualmente in via di trasformazione in carcere di massima sicurezza, e desta particolare preoccupazione il settore femminile, dove sono tuttora segregate 70 giovani donne, con 50 figli piccoli al seguito, detenute sulla base di processi svolti secondo il codice tribale. A tale proposito, sarebbe opportuno proporre la liberazione di queste detenute e l'affidamento del caso alla Commissione afghana sui diritti umani e a un collegio di giuristi che possa procedere alla loro riabilitazione, nonché al finanziamento di un programma di assistenza ad esse rivolto. Più in generale, è necessario fare il punto sulle condizioni di detenzione nelle varie carceri del Paese, per verificare se sono pienamente rispettati i diritti umani e gli *standard* internazionali. Altrettanto doveroso sarebbe rappresentare la preoccupazione del Governo italiano rispetto all'incolumità fisica della deputata Malalai Joya, di recente espulsa dal Parlamento afghano e ripetutamente minacciata di morte per le sue attività di denuncia delle responsabilità per le violazioni dei diritti umani nel Paese. Questa donna coraggiosa è un simbolo della resistenza delle donne afghane, fin da quando, in qualità di membro della Loya Jirga (l'Assemblea costituente del «nuovo Afghanistan»), denunciò i crimini dei signori della guerra che sedevano in quella stessa Assemblea. Più volte ospite nel nostro Paese, dove ha partecipato a vari incontri con parlamentari italiani, è oggi in una situazione di estremo pericolo e sarebbe grave se il nostro Governo non le esprimesse piena solidarietà per il suo operato e non si prodigasse per la sua sicurezza. Proprio il capitolo dei diritti umani merita, a mio avviso, una riflessione più ampia, soprattutto in relazione al tema della democrazia, per instaurare la quale, secondo la migliore tradizione delle nuove guerre, le truppe dell'Occidente occupano da tempo l'Afghanistan, l'Iraq e forse, un domani, l'Iran. Si tratta di "Stati canaglia", ci hanno insegnato, all'interno dei quali i diritti umani sono calpestati da dittatori sanguinari o da fanatici integralisti, che opprimono i loro popoli, li affamano e li privano di quel bene inestimabile, la democrazia, che potrebbe finalmente ripagarli delle tante sofferenze fin qui patite. Il problema è che questo bene supremo, la democrazia, per motivi misteriosi, o quantomeno non sufficientemente indagati, pare non riesca a germogliare autonomamente in queste terre, quasi che il DNA delle genti che vi risiedono ne fosse sprovvisto. Per rimediare a questa tara genetica, si è dunque pensato di importare i princìpi democratici da quei Paesi occidentali che ne dispongono in esubero e, come si fa con tutti i generi di conforto da destinare alle popolazioni affamate, si è scelto di farli piovere dal cielo, incapsulati in ordigni di vario genere. I primi esperimenti in questo senso risalgono alla guerra del Vietnam e sono documentati, oltre che dai libri di storia, da numerose testimonianze e reperti video messi a disposizione dagli stessi benefattori. Uno di questi documenti è stato realizzato, qualche tempo fa, in un servizio dell'emittente "Rainews 24": vi si ammira, nelle sequenze iniziali, una panoramica aerea della lussureggiante giungla vietnamita che, immediatamente dopo, riceve l'omaggio di una salvifica pioggia di napalm. Le bombe, ripiene di democrazia e *agent* *orange*, aprono squarci vermigli nel verde della vegetazione e, quando incontrano costruzioni, animali o esseri umani, li nebulizzano, trasformandoli, come per incanto, in sbuffi di vapore simili a quelli prodotti dai *geiser*. Questo suggestivo effetto visivo è ben documentato dalla telecamera piazzata sul ventre del bombardiere americano e ha per colonna sonora, realizzata dallo stesso ufficio propaganda dell'aviazione di quel Paese, una canzone di un gruppo musicale famoso in quegli anni, i "Mamas and Papas", intitolata "Sognando California", nella quale si vagheggia di grigi cieli invernali e di preti intenti nella preghiera. Non ho citato a caso questo documento: esso è infatti importante perché anticipa quella che diverrà una costante delle guerre moderne, e cioè la spaventosa percentuale di vittime civili, pari a circa il 90 per cento di quelle complessive. Erano civili i contadini vietnamiti polverizzati nelle loro capanne di giunchi mentre risuonavano le note dei Mamas and Papas; erano civili quelli che nel luglio del 2002 celebravano un matrimonio a Kandahar ed ebbero come inatteso regalo di nozze una bomba da 500 libre che uccise 100 di loro; erano civili, soprattutto bambini, quelli di un piccolo villaggio del deserto iracheno, Mogr-el-Deeb, sterminati l'anno successivo dagli elicotteri Apache. Sono civili almeno 80.000 vittime in Iraq dal 2003 e 63.000 in Afghanistan dal 2002. Una media di 62 morti al giorno, alla quale hanno contribuito, nelle ultime settimane, gli 87 uccisi dalle bombe NATO nella provincia di Oruzgan e a Kunjak, nel Sud dell'Afghanistan. Da sempre tali vittime sono state contabilizzate come «effetti collaterali», quasi che le nuove guerre fossero dei farmaci da sperimentare sul campo. Tuttavia, se un medicinale comporta cento di effetti indesiderati, lo si ritira immediatamente dal mercato, si apre un'inchiesta e si cerca di assicurare alla giustizia i criminali che lo hanno commercializzato. Perché, invece, gli effetti collaterali delle guerre, statisticamente assolutamente preponderanti, non inducono la benché minima riflessione sull'opportunità di proseguirle? Perché la guerra è l'unica strategia esentata dal fare i conti con la legge economica dei costi/benefìci? Eppure i dati parlano da soli: miliardi di dollari spesi in armamenti, centinaia di migliaia di morti, Paesi riportati all'età della pietra e, nonostante ciò, il benché minimo passo avanti fatto verso quella democrazia in nome della quale le guerre sono state scatenate. Ora, la Conferenza del 3 luglio viene indetta allo scopo di fare il punto sul sistema della giustizia in Afghanistan, il cui stato, tuttavia ci è ben noto. In particolare, ci è chiaro che in quel Paese c'è un gravissimo problema in materia di diritti umani e il primo e più importante dei diritti umani è quello alla vita, quotidianamente messo a repentaglio da azioni belliche che provocano vittime civili innocenti. Sarebbe assurdo non tenerne conto in sede di dibattito, così come sarebbe assurdo discutere della riforma del sistema giudiziario dimenticando che in Afghanistan c'è la guerra. Guerra e diritto, infatti, non vanno d'accordo: la guerra costituisce la negazione del diritto, si nutre delle sue ceneri. E il diritto non è una sfera simbolica fatta di formule e norme astratte, ma il riflesso di una società laddove essa sia libera di esprimersi. Al pari della democrazia non è importabile e, al di là di una serie di princìpi universali dei quali occorre esigere la rigorosa applicazione, esso si costituisce sulla specificità di un complesso sistema di usi, costumi e valori. Dunque, sarebbe bene tenere a mente il contesto in cui la Conferenza di Roma si inserisce: si tratta di un contesto emergenziale, dettato da una guerra in atto; non tenerne conto significherebbe celebrare una gigantesca rimozione. La Conferenza può essere comunque un'occasione per esigere la piena osservanza, da parte delle autorità afghane, dei diritti umani e delle convenzioni internazionali e per porre tale osservanza come condizione inderogabile per il prosieguo del rapporto di collaborazione tra i nostri Paesi; può essere la sede per ribadire che un processo di riconciliazione nazionale passa inevitabilmente attraverso il riconoscimento delle responsabilità di ciascuna delle parti in campo; può costituire un'opportunità concreta per dare vita a strumenti operativi, come, ad esempio, una commissione per la verità e la giustizia, in grado di far luce sulle violazioni dei diritti. Nondimeno, sono convinto che l'incontro di Roma si risolverebbe, comunque, in un'occasione mancata se non servisse a porsi delle domande sul futuro del nostro impegno in Afghanistan e sulla natura del rapporto che ci lega agli altri Stati "alleati". Al centro di questa apertura di dibattito, dovrebbe essere ovviamente il bilancio fallimentare segnato dalla strategia bellica e la necessità di riconoscere e riconsiderare scelte che si sono rivelate tragiche in primo luogo per la popolazione afghana. Se ci rendessimo protagonisti di un simile tentativo, potremmo ricollocare la questione del diritto e della giustizia nell'unico contesto che le compete, quello della costruzione della pace. Se, al contrario, alla Conferenza di Roma ci si limiterà a discutere di misure tecniche astratte, per loro natura inapplicabili in tempi di guerra, avremo perso l'ennesima occasione per prendere atto

Signor Presidente, signori del Governo, onorevoli colleghi, l'Italia ha assunto in Afghanistan un impegno molto importante, quello di coordinare le iniziative per la riforma della giustizia e dell'ordinamento giudiziario in quel Paese. Ebbene, le cose non vanno bene: nonostante l'impegno del Governo, non solo tutti gli elementi a nostra conoscenza ci dicono che questa riforma è molto indietro, ma il recente caso di Rahmatullah ha confermato che in quel Paese nessuna garanzia esiste, nemmeno del rispetto minimo dei diritti dell'uomo, persino quando si tratta di una persona prigioniera del Governo Karzai. Meritorio e positivo è stato l'impegno del Governo italiano per ottenere il risultato, ma non sfuggirà a nessuno che, se Rahmatullah è stato liberato, ciò è accaduto appunto per le pressioni del Governo italiano. Egli non ha avuto un giusto processo; non ha avuto un avvocato difensore; non è stato possibile conoscere i capi delle imputazioni; è stato nelle mani dei servizi segreti afghani contro persino quelle labili disposizioni di legge presenti in quel Paese. Abbiamo assunto un compito molto impegnativo, che non sarà facile svolgere. La Costituzione afghana, approvata nel gennaio 2004, un testo di elegantissima liberaldemocrazia, se non fosse che contiene un principio, all'articolo 3, in cui si afferma che in Afghanistan nessuna legge, Costituzione compresa, può essere contraria ai princìpi e ai precetti della sacra religione dell'Islam, e nel suo articolo 149, che corrisponde all'articolo 139 della nostra quella per cui la *sharia* prevale su qualunque altra legge, non è suscettibile nemmeno di revisione costituzionale. Allora, la verità è che, in questo momento, il Governo difeso dagli occidentali e la zona di territorio da esso governata sono soggetti alla *sharia*, alla legge islamica, alla legge islamica, come fonte prevalente su ogni altra. Se questo certamente non fa piacere quando accade in Paesi che sono considerati nemici dell'Occidente, non ci dobbiamo nemmeno nascondere che ciò accade per solenne proclamazione della Costituzione afghana, in quel Paese, del quale noi, in teoria, saremmo chiamati a difendere la democrazia rispetto agli attacchi dei nemici della medesima. Particolarmente grave è la violazione dei diritti umani che riguardano le donne. Siamo arrivati al punto, sempre in applicazione della *sharia*, che la deputata Malalai Joya è stata addirittura espulsa dal Parlamento afghano per aver osato presentarsi in quella sede in vesti, in forme e con un linguaggio non sottomessi alla primazia patriarcale maschile di quel sistema ed è continuamente minacciata di morte. È questa la democrazia che stiamo difendendo? Sono questi i diritti umani che stiamo difendendo? È per questo che c'è stato un intervento militare al termine del quale, con grande retorica, si disse che le donne afghane erano finalmente liberate dall'oppressione islamica?

Forse non ci turbiamo perché quegli uomini, donne e bambini sono di un'etnia, una pelle o una fede religiosa diverse dalle nostre, ma la verità è che le forze da noi sostenute stanno procedendo, secondo la spietata logica della guerra del nuovo millennio, con bombardamenti indiscriminati e che causano vittime civili, e ciò davvero colpisce la sensibilità etica di tutti noi. La verità è - e qui passiamo dalle considerazioni etiche e costituzionali, pur rilevanti, alla politica, perché non risulta essere stata abrogata la norma costituzionale che vieta il ricorso alla guerra come mezzo di risoluzione dei conflitti internazionali - che alcuni alcuni di noi, fin dall'inizio del massiccio impegno militare italiano in Afghanistan, dichiararono la loro contrarietà. Per disciplina di maggioranza abbiamo votato le decisioni di continuità del Governo di centro-sinistra, ma la verità è che purtroppo avevamo ragione; purtroppo, eravamo profeti: la guerra in Afghanistan si sta rivelando non già uno strumento di esportazione della democrazia e dei diritti umani, di difesa della libertà, ma una nuova forma, praticamente indistinguibile rispetto all'Iraq, della guerra al terrorismo dichiarata dall'Amministrazione Bush. Questa guerra, guerra, non solo per i nostri princìpi, ma anche per considerazioni di realismo politico, è profondamente sbagliata. In primo luogo, essa crea basi territoriali ad Al Qaeda. In Iraq c'era Saddam Hussein, certamente un pericoloso dittatore; adesso, non solo c'è una guerra civile in corso, ma c'è una base territoriale per i fondamentalisti di Al Qaeda, che si stanno spostando anche in altre parti del mondo islamico, dalla Somalia al Libano e, speriamo di no, anche alla Palestina. Questo tipo di guerra indiscriminata, senza regole e rispetto del diritto internazionale, sta alimentando il terrorismo. Il nemico al quale la guerra era stata dichiarata, purtroppo, rischia di vincerla per effetto della guerra medesima. La guerra è sbagliata anche per una seconda ragione, che rende di fondamentale importanza, da parte nostra, la scrupolosa attenzione a che non siano violati i diritti umani, particolarmente per l'Italia, particolarmente nel territorio controllato dal Governo Karzai e particolarmente perché abbiamo assunto l'impegno di rinnovare il sistema giudiziario di quel Paese. Paese. L'Occidente, infatti, si mostra, davanti al mondo islamico, come il mondo ipocrita della doppia verità. Guantanamo, Abu Ghraib, le torture, la violazione dei diritti umani perpetrati perpetrati dall'Occidente vengono percepiti nel mondo islamico come l'ipocrisia di chi pretende di esportare la democrazia e i diritti ed è il primo a violarli. Non è un caso che, in tutti i Paesi islamici dove si vota liberamente, si stanno affermando non le forze laiche, che pure esistevano in questo Paese, ma forze legate, in maggiore o minore misura, al fondamentalismo islamico. È la reazione di un mondo intero che non si identifica nel terrorismo (sono noti i contrasti, per esempio, fra Hezbollah, Hamas e persino Fratellanza musulmana, in Egitto, e Al Qaeda), ma assume una propria identità islamica, profondamente sbagliata e pericolosa, come reazione alla doppia morale di un Occidente che appare loro ipocrita e voglioso solamente di potenza. Come si vede, la politica della pace non è massimalismo, non è radicalismo, ma è oggi l'unica politica realistica. Ripetiamo, non è seguendo le scelte dell'Amministrazione Bush sempre più contestata, del resto, sia negli Stati Uniti d'America (come risulta dalle recenti elezioni congressuali, dove è prevalso il partito democratico, che assume una linea politica diversa), sia nell'altro Paese che l'ha condivisa.

Occorrerà tornare a discuterne, ma intanto abbiamo ritenuto giusto - e confidiamo che il nostro Governo faccia questo - impegnarsi davvero e fino in fondo per la protezione dei diritti umani lì dove abbiamo la possibilità di farlo, come oggi a Kabul. a Kabul. Non è tutto, ma non è poco. Mostriamo l'altro volto dell'Occidente. L'Italia è in grado di farlo per le sue tradizioni democratiche, per i suoi princìpi costituzionali. Mostriamolo, però, signori del Governo, davvero e fino in fondo, senza impantanarci nella *realpolitik*, altrimenti l'Occidente, per la responsabilità di chi segue apparentemente una logica di *realpolitik*, ma che in realtà è fallimentare, si troverà davvero in difficoltà e senza difese di fronte all'offensiva che proviene dal resto del mondo.

rappresenta ancora una volta la fotografia delle diverse anime della maggioranza e, in alcune parti, la grave contrapposizione che divide e dividerà fino alla caduta di questo Governo le varie componenti politiche della maggioranza. In molti argomenti la maggioranza è divisa, ma ancor più è divisa su un argomento così scottante come quello dell'Afghanistan. Se da noi oggettivamente può essere condivisibile qualche generica affermazione di principio sulla giustizia, certamente è da respingere, anzi da riprovare, tutta la parte sostanziale del testo, che a noi sembra una vera e propria provocazione. Si ringrazia infatti il Governo per aver provocato una straordinaria mobilitazione dell'opinione pubblica internazionale per il proscioglimento di Rahmatullah Hanefi, per aver costui svolto un ruolo indispensabile di mediazione per la liberazione del giornalista de «la Repubblica», Daniele Mastrogiacomo, e di Gabriele Torsello. A parte le considerazioni squisitamente umane sull'intera vicenda, come possiamo associarci al ringraziamento rivolto ad un Governo che con il proprio operato

un'ombra nera sulla sua politica estera e procurandole seri attacchi da parte dei suoi alleati americani e, ancor più, della Germania che, con durissime parole della stessa Merkel, ha criticato il suo operato?

di giustizia umanitaria, oltre che penitenziaria, in relazione alle disumane situazioni in cui oggi versa tutta la popolazione civile dell'Afghanistan. Ma com'è possibile, signor Presidente, considerare un Paese di civiltà quello in cui si tengono recluse donne con i propri bambini? Questo è il vero punto fondamentale di cui ci dobbiamo occupare e sul quale possiamo certamente dare un contributo forte con le nostre mozioni.

Signor Presidente, onorevole rappresentante del Governo, onorevoli colleghi, esprimo un grande rammarico ed una seria preoccupazione. Il rammarico è per il fatto che un tema di questa straordinaria importanza come abbiamo ascoltato fino ad ora - sostanzialmente non veda impegnato il Senato della Repubblica con la stessa intensità con la quale esso è impegnato in altre circostanze. La preoccupazione consiste nel fatto che questa vicenda, occasionata da una mozione presentata da alcuni colleghi del centro-sinistra - nel testo originario,

si affronta il tema dell'imminente Conferenza internazionale sulla giustizia in Afghanistan, promossa dall'Italia, per discutere più generalmente della questione riguardante L'UDC non ha nulla in contrario a che si discuta in via generale della questione dell'Afghanistan, come della politica estera del Governo Prodi e del possibile segretario generale del Partito Democratico Veltroni, il quale, per la verità, ieri non ha fatto alcun accenno alla politica estera del nostro Paese. Non ho capito se il voltar pagina significhi, per esempio, cambiare anche la politica estera o meno. Non so se la nuova Italia di cui parla Veltroni sia un'Italia della quale non debbano far parte quelli che ci sono stati fino ad ora o altro. Non lo so, sta di fatto che nel non breve intervento dell'onorevole Veltroni a Torino non vi è stato un solo passaggio, dico un solo passaggio - ho avuto la fortuna di poterlo ascoltare integralmente - dedicato alla politica estera. Mi chiedo cosa significhi questo fatto. Quindi, signor Presidente, mi permetto, dando pure dando pure per scontato che l'onorevole Veltroni può conoscere gli atti del Senato senza alcuna difficoltà acquisendoli, di chiedere formalmente che gli vengano trasmessi gli atti della discussione che si sta svolgendo oggi in quest'Aula sul tema della giustizia in Afghanistan

di una Conferenza internazionale sulla giustizia in Afghanistan in totale continuità con il Governo Berlusconi, che è all'origine dell'impegno particolare che le Nazioni Unite hanno affidato all'Italia di promuovere la ricostruzione dell'ordinamento giudiziario afghano sulla base di una decisione assunta nel 2001. Tale decisione nacque, ovviamente, non per una generica volontà di potenza dell'Occidente nei confronti degli sventurati afgani, ma come risposta, che all'epoca fu ritenuta unanime da parte di tutto il mondo occidentale e orientale, all'indomani di un attentato molto sanguinoso, con più di 2.000 morti, provocato negli Stati Uniti, che in qualche misura dobbiamo riportare al centro della nostra attenzione, altrimenti non si capisce di cosa stiamo parlando. Confermo quindi la richiesta che vengano trasmessi all'onorevole Veltroni i documenti, gli atti, le mozioni, gli interventi e tutto ciò che è pubblico perché è opportuno che se ne faccia una motivazione particolare. Da questo punto di vista, l'UDC è interessato a porre in evidenza una considerazione: all'Italia fu affidato, per decisione delle Nazioni Unite, non dell'Amministrazione Bush, un compito di straordinario rilievo culturale, giuridico e politico, quello di procedere alla costruzione dell'ordinamento giudiziario afghano,

lo erano sistematicamente. L'UDC dà per scontato che non esista una politica internazionale che possa procedere alla costruzione di un ordinamento giudiziario senza un'adeguata tutela dei diritti umani in quell'ordinamento quindi, concordiamo assolutamente con chi ha voluto affermare, in quest'Aula o nelle mozioni presentate, il presupposto della rigorosa tutela dei diritti umani perché si possa parlare di un ordinamento giudiziario degno di questo nome.

parte, ma il Governo italiano dal dicembre 2001 fino ad oggi, in ordine alla costruzione dell'ordinamento giudiziario afghano. Lo dico perché ho avuto l'impressione che non se ne parlasse quasi più. Occorre invece capire che questo era, ed è, l'oggetto principale della Conferenza internazionale, ed è la ragione per la quale il Gruppo UDC concorda totalmente con la mozione Calderoli-Castelli, la prima delle tre, perché ripercorre tutta la trama, per così dire, degli interventi affidati all'Italia a partire dal dicembre 2001, con particolare riferimento a ciò che è stato fatto nel corso di cinque anni, dal 2002 in poi, dal Governo italiano in Afghanistan su questa vicenda. La domanda è se è stato fatto qualcosa o no, sono stati approvati i codici civile e penale, di procedura civile e penale. La risposta è sì e allora mi sembra innanzitutto doveroso che il Senato della Repubblica esprima apprezzamento al Governo italiano nella sua completezza, Governo del passato e Governo attuale, in totale continuità. Possiamo dire che siamo insensibili ai problemi della difesa dei diritti umani? No, non siamo insensibili. Possiamo ritenere che vi siano tuttora carenze gravi in ordine alla tutela dei diritti umani in Afghanistan? Riteniamo che questo possa essere il caso e che quindi il Governo italiano debba riferire sul modo in cui la tutela dei diritti umani è stata soddisfatta fino ad un certo punto e non è soddisfatta in altri punti, partendo anche dalla considerazione della vicenda Hanefi. Ci mancherebbe altro. Abbiamo espresso la nostra soddisfazione particolare per il fatto che si sia ritenuto che Hanefi non fosse responsabile di reati particolari, ma non è che ci sia un processo Hanefi come unica questione posta in Afghanistan. Non c'è un problema delle carceri speciali afghane come il problema delle carceri speciali. L'Italia non ha finanziato carceri speciali in Afghanistan, né con il Governo Berlusconi, né con il Governo Prodi. Occorre che sia chiaro capire, da questo punto di vista, che noi stiamo operando in un territorio che aveva le carceri speciali, aveva la violazione dei diritti umani come origine ed era il Governo talebano. Da questo punta di vista, non stiamo operando in un Paese nel quale fioriva, prima del nostro intervento, la regola del diritto, la *rule of law*, come dicono gli americani: era un Paese nel quale occorreva costruire i presupposti di ciò e e quindi il giudizio politico che vogliamo esprimere è anzitutto su ciò che è stato fatto in questa specifica vicenda. Perché all'Italia è stato assegnato questo compito? Da chi è stato assegnato? Qual è l'obiettivo strategico di questo compito? È stato assegnato dalle Nazioni unite all'indomani dell'attacco alle Torri gemelle, non per una volontà di potenza imperiale, ma per una volontà di ripristino dell'ordine internazionale violato. Si tratta di capire che queste sono le questioni fondamentali: il ripristino dell'ordine internazionale violato. Non c'è una scelta tra pace e guerra, come pure è stato detto. Credo che se mettessimo la questione a *referendum* saremmo tutti per la pace; non credo che nessuno possa essere per la guerra, in questo Parlamento. Ovviamente, sappiamo che la pace è un obiettivo strategico, non è un punto al quale tendere senza alcuna condizione. Non voglio ricordare ancora una volta, come spesso si dice, che se avessimo scelto la pace anziché la guerra avremmo ancora, probabilmente, Mussolini ed Hitler. Il dato di fatto non è la questione di chi sia il nemico in quel momento, ma la questione che lo strumento della rinuncia all'uso delle armi è di per sé inidoneo a garantire la sicurezza,

perché è il sindaco della città di Roma, che come tale è il cuore della politica internazionale del Paese. Forse lo ha fatto perché sa che all'interno della maggioranza che dice di voler sostenere vi sono due opinioni di politica estera Può darsi che non abbia voluto parlare perché è consapevole che sulla politica estera si gioca la sostanza del Partito democratico e del Governo Prodi. Questo è ciò che è emerso nel dibattito, nel quale ho l'impressione che il tema dell'ordinamento giudiziario afghano sia stato utilizzato più come occasione per un dibattito generale sull'Afghanistan che come argomento specifico strategico. È questa la ragione per la quale, signor Presidente (lo dico all'onorevole Angius, un attimo fa l'avevo chiesto al collega Calderoli), ribadisco che, per quanto riguarda l'UDC, riteniamo opportuno che vengano trasmessi all'onorevole Veltroni tutti gli atti che riguardano il dibattito di politica estera di oggi al Senato

l'onorevole Veltroni si possa rendere conto del fatto che l'ordinamento giudiziario afghano è stato affidato all'Italia, come Paese guida, nel 2001, non nel 2007, e che occorre esprimere un giudizio su ciò che il Governo italiano ha fatto in questi cinque anni e non soltanto in questi ultimi mesi.

Sono queste, signor Presidente, le ragioni per le quali un dibattito generale sulla politica estera del Paese si è svolto in occasione dei decreti-legge che hanno riguardato il rinnovo o l'ampliamento del finanziamento italiano alle missioni internazionali. Non abbiamo difficoltà a ripetere un dibattito generale sulla politica estera, compresa quella in Afghanistan. Non abbiamo alcuna difficoltà a poter mettere in evidenza il risultato che si ottiene in Afghanistan rispetto a quello dell'Iraq. Vogliamo soltanto far presente che in Afghanistan non siamo stati mai in presenza di una volontà di potenza degli Stati Uniti nei confronti di quel Paese, siamo stati in presenza di una risposta delle Nazioni Unite ad una violazione della legalità internazionale compiuta attraverso l'attentato alle Torri gemelle. Questa distinzione, che poi rappresenta la continuità totale della politica estera italiana, mi sembra importante perché è nell'ambito di questa continuità

devo dirle - come lei ben sa - che gli atti sono pubblici. L'onorevole Veltroni per ora è sindaco di Roma, so benissimo, come lei, che si è candidato alla guida del futuro Partito democratico; per una questione di *par condicio*, direi di inviare gli atti anche a tutti gli altri possibili candidati alla guida del Partito democratico. Signor Presidente, onorevoli colleghe e colleghi, se volessimo cercare esempi viventi delle contraddizioni, dei ritardi e della drammaticità della situazione Il primo è quello di Malalai Joya, giovanissima deputata del nuovo Parlamento afghano. Chi, come me, ha avuto occasione di conoscerla personalmente, come molte altre donne parlamentari del Gruppo di contatto, non può non rimanere impressionato dal coraggio civile e dalla determinazione che Malalai mette nel suo atto costante di denuncia delle violazioni dei diritti umani del Paese commesse dai talebani e dai signori della guerra. Lei, e migliaia di altri afghani, hanno guardato con sentimenti contrastanti e contraddittori alla presenza militare straniera, sperando che questa portasse perlomeno ad una cesura netta con la storia passata, quella appunto dei talebani e dei signori della guerra. A loro oggi resta solo l'amarezza di vederli saldi nei loro scranni in Parlamento e nel Governo Karzai. E così Malalai oggi viene espulsa dal Parlamento, dopo essere stata oggetto di continue minacce di morte da parte di suoi stessi colleghi parlamentari, una situazione inaccettabile che a nostro parere richiede l'immediata attivazione da parte del Governo italiano per un suo immediato reintegro in Parlamento. Il secondo caso è quello Rahmatullah Hanefi, il mediatore di Emergency detenuto senza imputazione - come è stato giustamente sottolineato dal senatore Salvi - per aver lavorato su richiesta esplicita del Governo italiano alla liberazione di Daniele Mastrogiacomo. Una storia a lieto fine, quella di Hanefi, di recente liberato, ma che a nostro parere rende bene il quadro nel quale oggi si sviluppa il sistema giudiziario in Afghanistan: un sistema ancora "balcanizzato", ispirato a ben tre codici, a leggi tribali, alla Sharia, che si intreccia con le ossessioni securitarie e le eccezioni che gli Stati Uniti d'America vorrebbero introdurre in ossequio alla loro crociata contro il terrorismo. L'Afghanistan Compact, al quale l'Italia si è impegnata a livello di *Joint Coordination and Monitoring Board* (JCMB) e anche come *lead country* per quanto riguarda le riforme nel settore della giustizia, accanto alla componente militare a quella della ricostruzione, aveva delineato un programma di lavoro per la riforma al settore, per la *rule of law*, per i diritti umani, tuttora bloccato nelle commissioni miste competenti. Vorrei ricordare che l'Afghanistan Compact si regge su tre piedi: quello della giustizia, della *rule of law* e della democrazia; quello della ricostruzione fisica delle fisica delle infrastrutture e la lotta alla povertà; quello della sicurezza intesa principalmente come attività militare del contingente ISAF. Di questi tre piedi, due oggi non funzionano, sia quello militare, come avrò occasione di dimostrare, sia quello della ricostruzione civile. Il problema, quindi, oggi non è soltanto procedurale, ma anche di sostanza politica. Se vogliamo parlare di giustizia economica, ad esempio, quale giustizia economica ci può essere in un Paese dove il 70 per cento della popolazione oggi è malnutrito e non può accedere al cibo? Se parliamo di giustizia e legalità, legalità, questo stallo inaccettabile rafforza il potere dei signori locali, indebolisce il già debole Governo Karzai e soprattutto sottopone centinaia di donne e uomini afghani a vessazioni ed inaccettabili violazioni dei loro diritti fondamentali. Il Paese vive ancora nell'impunità dei crimini attuali e di quelli pregressi. Il piano di giustizia transizionale approvato dal Governo Karzai nel 2005 è ancora in gran parte inapplicato, soprattutto per quanto riguarda il perseguimento delle violazioni dei diritti umani compiute prima, durante e dopo la caduta del regime talebano. È per questo motivo che chiediamo e pensiamo che questo sia un elemento fondamentale per garantire coerenza rispetto a quello che il Governo italiano dice di voler fare in Afghanistan sui diritti umani, sul buongoverno e sulla democrazia. Alcuni, come RAWA ed altre organizzazioni afghane, chiedono la creazione di un tribunale internazionale che possa giudicare i crimini commessi dai signori della guerra, dai talebani e non solo. Pensiamo che questa possa essere una importante opportunità da analizzare e da elaborare in maniera più coerente e cogente. Come denuncia Amnesty International nel suo ultimo rapporto annuale, anche molti governatori locali continuano ad operare in assoluta autonomia dal Governo centrale continuano a violare gravemente i diritti umani. Le forze di sicurezza afgane, in particolare la polizia, continuano a detenere illegalmente i cittadini afghani e a torturarli. Centinaia sono le donne detenute in condizioni indecenti in seguito a condanne comminate secondo i codici tribali, per adulterio o reati affini. un aumento dei casi di delitti d'onore e anche di autoimmolazione delle donne in una società che rimane brutalmente patriarcale al punto che le stesse donne subiscono violenza anche dai giudici e dai poliziotti che dovrebbero tutelarne i diritti. Poi c'è il carcere di Pol-i-Chark, finanziato anche dal Governo italiano, dove oggi 70 donne e 50 bambini vivono in condizioni inumane e indecenti. Questa struttura, un penitenziario civile, verrà trasformata in un penitenziario di massima sicurezza e ospiterà anche i detenuti che provengono da Guantanamo e da altre basi militari americane in Afghanistan, come quella di Bagram, dove attualmente sono 500 detenuti in attesa di giudizio. Cosa pensiamo noi, cosa pensa il Governo italiano rispetto a questa situazione e rispetto alle legislazioni di emergenza che gli americani continuano ad applicare e ad imporre anche sulle popolazioni civili afgane? Il Governo è perfettamente consapevole della situazione; riteniamo debba cogliere l'occasione della Conferenza internazionale per chiedere la liberazione di quelle donne e la loro riabilitazione e programmi di reinserimento e di supporto per quelle famiglie già duramente provate. Malalai, Hanefi, le detenute di Pol-i-Chark e tutto il popolo afghano oggi sono presi nel mezzo di un conflitto sempre più aspro, di una realtà quotidiana nella quale lo stesso concetto di giustizia scompare miseramente. Da una parte, i talebani non esitano ad assaltare scuole e villaggi e seguono una politica deliberata di uccisione di civili. le operazioni militari della NATO e di *Enduring freedom* mietono vittime civili, danni collaterali di bombardamenti indiscriminati. C'è un punto sul quale vorrei richiamare l'attenzione di tutti: le forze internazionali ISAF oggi godono di uno *status* legale che le pone al di là della legge afghana e anche al di là delle nostre normative nazionali; lo dice Amnesty International. Questa situazione di fatto comporta una sorta di esenzione delle truppe internazionali da ogni forma di responsabilità nei confronti del diritto internazionale. Quindi, i bombardamenti ISAF possono svolgersi violando il diritto internazionale umanitario e anche le nostre truppe rischiano di farlo quando consegnano alle autorità afgane o a quelle americani i prigionieri, senza poter accertare se poi questi vengono o meno sottoposti a tortura. Questi sono elementi importanti che evidenziano la necessità di una maggiore coerenza nell'impegno per i diritti umani in quel Paese. Il ministro Parisi, di recente, ha giustamente denunciato le vittime civili causate dall'operazione ISAF. Questo, però, non basta: noi chiediamo che venga costituito un organismo al quale le popolazioni civili possano ricorrere per chiedere certezza sulle responsabilità di quelle vittime ed un risarcimento equo ed immediato.

che l'unica via d'uscita dal disastro causato dall'avventura militare afghana sia quella della ricostruzione del tessuto sociale ed economico, della convivenza civile, della riattivazione delle reti di società civile dal basso, di democrazia vera e non formale, dei diritti umani e della fine dell'impunità. Per tale motivo, chiediamo anche che l'Italia si impegni, e colga l'occasione della Conferenza internazionale sulla giustizia per farlo, in una rimodulazione della presenza internazionale in Afghanistan. Non vogliamo lasciare il popolo afghano in mano ai talebani, ai signori della guerra o ai contingenti americani *Enduring freedom*;

utilizzare l'occasione della Conferenza internazionale sulla giustizia per trarre quegli elementi necessari per costruire quella Conferenza internazionale sull'Afghanistan della quale abbiamo perso traccia nella stampa e nelle dichiarazioni pubbliche del Governo stesso ed anche a rivedere il mandato delle truppe ISAF affinché vengano sostituite con un contingente internazionale di polizia sotto l'ombrello dell'ONU. Lo sta già facendo l'Europa con la missione PESD, inviando civili, cioè poliziotti, avvocati avvocati ed osservatori sui diritti umani. Pensiamo che questa debba essere la strada da perseguire e che si debba fare presto. L'Italia, infatti, ad ottobre dovrà riferire al Consiglio di sicurezza dell'ONU sull'ISAF e riteniamo che questa scadenza non possa essere mancata. Solo a queste condizioni, onorevoli colleghe e colleghi, pensiamo che la Conferenza sulla giustizia possa avere un senso e non rischi di diventare un evento autocelebrativo. Per questo sosterremo con il nostro voto favorevole la mozione n. 115 (testo 2), da noi presentata, impegnandoci però ad intensificare il lavoro e gli sforzi

i legami tra sicurezza, sviluppo e giustizia e promozione e tutela dei diritti umani sono inscindibili. Questo convincimento ha indotto la comunità internazionale ad affrontare i temi nella Conferenza di Bonn del 2001, nella quale sono state stabilite le tappe del processo di ricostruzione politica e statuale dell'Afghanistan; con la successiva Conferenza di Tokyo del 2002 si è delineato il percorso della ricostruzione delle istituzioni statutarie afgane con il sostegno - appunto - della comunità internazionale. Per quel percorso, all'Italia fu affidato il ruolo di Paese *leader* per la riforma della giustizia: si è trattato pluriennale, finalizzato alla costruzione giuridica, nel rispetto degli *standard* internazionali ed anche dei diritti umani. È stato un compito veramente impegnativo, se si valuta in un contesto istituzionale, politico ed anche consuetudinario della giustizia. Infatti, la costituzione materiale del diritto in Afghanistan è basata, per la stragrande maggioranza dei casi, su codici tribali e sulla stessa *sharia*; tali consuetudini prevalgono e la maggior parte delle incriminazioni e delle sentenze che portano ad una pena e ad una detenzione risponde ancora alla logica dei codici tribali. Lo raccontava il rappresentante dell'Unione Europea Vendrell quando affermava che l'Italia partecipa attivamente alla riforma del sistema giudiziario e sottolineava il fatto che il processo costituente rappresenta la parte facile o meno difficile, mentre risulta complicato ripristinare lo Stato di diritto, riformare le forze di polizia e costruire un sistema giudiziario. In Afghanistan - ricordava esistono tre diversi sistemi giuridici: il diritto civile, la legge islamica e il diritto consuetudinario. l'approvazione della nuova Costituzione e la Conferenza di Londra del gennaio 2006, che con il piano "*Afghanistan* *Compact*" definì gli aiuti economici e il documento politico quinquennale che traccia le linee guida

istituzionali e statuali. Aggiungasi che nel corso del 2005, mentre continuava il nostro impegno finanziario, si è complicato il sistema di collaborazione tra il nostro Ufficio italiano giustizia, la struttura che costituiva la gestione del programma di giustizia in Afghanistan, e il sistema più complesso delle Nazioni Unite, secondo quanto stabilito nella Conferenza di Londra. Pertanto, l'Ufficio italiano giustizia un po' ridimensionato o, comunque, molto più complicato il proprio ruolo basato antecedentemente su un rapporto bilaterale. Si è pertanto innescata una problematica più complessa di gestione attraverso un'applicazione trilaterale (agenzia ONU, Italia, istituzioni afgane) che ha ricondotto la nostra funzione ad una *partnership* trilaterale. Questi problemi non devono distoglierci; devono anche essere di pungolo per continuare la nostra azione volta a migliorare il sistema giuridico afghano. Infatti, la riforma varata ha introdotto concetti giuridici innovativi, soprattutto se li valutiamo applicati ai minori e alle donne; la riforma penitenziaria attraverso strutture operative deve essere completata per intercettare abusi e maltrattamenti. È necessario un maggior coinvolgimento di giustizia per promuovere la corretta diffusione della riforma legislativa; è urgente una serie di iniziative finalizzate al recupero, alla formazione al reinserimento socio-economico dei minori detenuti. Quindi, molto c'è da fare ancora, e da questo punto di vista, come sosteneva il rappresentante delle Nazioni Unite, grazie all'aiuto italiano siamo di fronte ad un sistema giudiziario in via di formazione; non è ancora perfetto, sono necessari molti miglioramenti, ma sono in corso processi in cui gli avvocati già garantiscono la difesa degli imputati. È in questo contesto che l'ordine del giorno G1 intende

Signor Presidente, quello che stiamo svolgendo è un dibattito difficile da seguire perché ogni orattore interviene con una sfaccettatura e un aspetto particolare,

giudiziario afghano, programmata dal 3 al 7 luglio, è stata rinviata più volte, e più volte si è detto che tale Conferenza era inserita all'interno di un ragionamento che riguardava anche la liberazione degli ostaggi. Non credo sia difficile immaginare che per i talebani una Conferenza sulla riforma della giustizia in Afghanistan non sia propriamente argomento di grande interesse, ma nello stesso tempo questa Conferenza - e il senatore Tonini lo ha in parte riconosciuto - dal Governo italiano veniva caricata di una valenza che va al di là

pace. La prima considerazione è che il contenuto della Conferenza non è affatto in discussione in quest'Aula, perché francamente credo interessi molto poco, e forse solamente a qualche addetto ai lavori. Ha invece una valenza politica, e qui si spiega anche la mozione Salvi, almeno la mozione Salvi che tentava, di fronte alla scadenza del 3 luglio, di aprire un dibattito all'interno del Parlamento, ma credo soprattutto all'interno della maggioranza,

se dobbiamo parlare di Afghanistan e della spedizione in Afghanistan, ci sono momenti e sedi opportune nelle quali possiamo discutere dell'aspetto militare, della ricostruzione civile, dei piani di ricostruzione provinciali, della riforma della giustizia. Se vogliamo parlare di riforma della giustizia in Afghanistan, lo possiamo fare; ne parliamo solo per capire se, da quando nel 2002 il Governo di allora si assunse, su invito delle Nazioni Unite, l'onere della riforma della giustizia, questo Governo e i nostri funzionari sul terreno hanno ben operato, se qualche cambiamento all'interno di una struttura, collega Martone, che non è quella di una ex democrazia passata per due o tre anni, provvisoriamente, nel regime talebano, ma che è radicata nella storia tribale dell'Afghanistan che credo tutti conoscano. Per questo, sentendo oggi alcune affermazioni, peraltro assolutamente legittime e in teoria condivisibili del senatore Martone, applicate all'Afghanistan, mi sembra di ragionare su due piani profondamente diversi. Certamente, è difficile immaginare che in due o tre anni il *burqa* possa sparire dall'Afghanistan: credo che chi è stato anche recentemente a Kabul abbia visto come questo fenomeno, abbastanza visibile,

e alleati. Se questo era il problema politico, evidentemente si è svolto un dibattito non in quest'Aula, ma in altre sedi assolutamente legittime, nei corridoi e negli uffici, per ricompattare una maggioranza attorno ad un discorso che evidentemente, ponendo in discussione l'Afghanistan, denota la debolezza della maggioranza a reggere sia l'interevento militare, sia la ricostruzione civile, sia la ricostruzione della giustizia e l'impegno complessivo che noi abbiamo tenuto, mantenuto ed anche - per dichiarazione del ministro Parisi - che continueremo a mantenere secondo il Ministro per molti anni, rispetto alla vicenda afghana che evidentemente ad una parte della maggioranza non interessa, almeno nella misura in cui noi la presentiamo. Questo andava detto nel dibattito di oggi, se volevamo essere coerenti, anche per inquadrare all'interno di una missione strategico-politica questa Conferenza sulla giustizia che altrimenti - mi rendo conto com'è nata e per come doveva essere, è semplicemente una conferenza di tecnici, di esperti che vanno a valutare quanto noi abbiamo proposto. E abbiamo proposto molto: ci sono le riforme dei codici; certo non sono ancora applicate, ma questo è uno dei temi che la Conferenza deve affrontare per capire le ragioni di un ritardo che indubbiamente esiste, degli ostacoli che devono essere risolti, che non sono solo di Karzai, ma della realtà di questa benedetta società civile afghana. Una società che indubbiamente, nella sua minoranza

- anche voi avete accennato a questo - su che senso ha una democrazia in un Paese, se il linguaggio che è alla base della stessa democrazia non è quello comune e non è il sistema dei valori condivisi.

Noi possiamo insegnare delle tecniche, che è quel che stiamo cercando di fare sulla riforma della giustizia. Possiamo insegnare o portare, come abbiamo fatto in molti casi, delle tecniche parlamentari, ma non credo si possa assumere l'atteggiamento che è stato assunto in quest'Aula.

la guerra al terrorismo si fa cercando di capire o di accettare che Hamas ed Hezbollah siano due movimenti politici. Vorrei capire se la guerra al terrorismo si fa cercando di capire le ragioni di Al Qaeda,

Vorrei capire se siete tutti per il Governo di unità palestinese per ridare il tempo ad Hamas di organizzarsi e conquistare Gaza, non con una guerra civile, ma con esecuzioni programmate e progettate da Hamas con gente buttata dal decimo piano dei palazzi di Fatah.

È quella di non capire che non esiste una fratellanza araba e una posizione politica congiunta e comune del mondo arabo che possa aiutare anche noi ad affrontare questi problemi? Come si fa sul piano politico, secondo voi? Continuate a lamentarvi senza

che tengano conto delle realtà che esistono sul terreno, per cui bisogna andare da Hezbollah e da Hamas a spiegare che il dibattito si fa in Parlamento e non con le mitragliatrici e con i razzi, e che magari, per essere accettati nella comunità internazionale, bisogna anche dichiarare che Israele ha il diritto di sopravvivere, cosa che non mi pare che Hamas ed Hezbollah abbiano ancora fatto. Venendo al tema oggetto della nostra trattazione, mi sembra che sulla Conferenza internazionale della giustizia non ci sia altro da aggiungere; è un fatto tecnico. Noi abbiamo presentato

Signor Presidente, signori rappresentanti del Governo, onorevoli colleghe e colleghi, democrazia e protezione dei diritti umani rappresentano le fondamenta di un progresso sostenibile e politico di tutti i Paesi e quindi, in modo particolare, per l'Afghanistan, il cui Governo è chiamato a dare priorità alla creazione in ogni provincia di istituzioni funzionanti quali l'amministrazione civile, la polizia e il sistema giudiziario. L'obiettivo del sistema giudiziario è garantire un accesso alla giustizia equo e trasparente, basato su codici scritti, giusti processi e verdetti esecutivi. I punti relativi a «*governance* e diritti umani» sono la riforma della pubblica amministrazione, la lotta alla corruzione, i censimenti e statistiche, le assemblee nazionali, le elezioni, la parità sessuale, lo Stato di diritto, le registrazioni delle terre e la lotta ai narcotici e ai diritti umani. Già durante il dibattito sulla missione in Afghanistan qui in Senato, le colleghe di tutti gli schieramenti hanno ottenuto un importante risultato: l'approvazione dell'ordine del giorno che impegnava il Governo a promuovere e sostenere un'azione, tesa ad intensificare i contatti tra le donne rappresentanti del Parlamento italiano e le donne rappresentanti le istituzioni e la società civile afghana. Questa è la strada che vogliamo continuare a percorrere, cari colleghi. Gli Accordi di Bonn del dicembre 2001 e la Conferenza di Tokyo del 2002 hanno fissato i princìpi per la ricostruzione delle istituzioni statutarie afgane e l'Italia. In questa circostanza, ha assunto un ruolo *leader* con un programma di giustizia pluriennale, attraverso il ripristino dell'amministrazione giudiziaria in linea con gli *standard* internazionali sui diritti umani, e qui va ricordato, grazie al Governo Berlusconi. Tuttavia, prevalgono ancora i codici tribali rispetto all'applicazione della giustizia di uno Stato di diritto e per questo l'Italia si è impegnata, coinvolgendo le organizzazioni internazionali, nella realizzazione di questo programma di giustizia. Si è arrivati, quindi, alla predisposizione di un pacchetto di riforme legislative, su cui la comunità internazionale e il nuovo Parlamento afghano hanno potuto operare. Tale riforma della giustizia ha introdotto aspetti innovativi a favore dei minori e delle donne e questo è già una prima conquista. Dobbiamo continuare su questa strada. Molto si è fatto, molto è ancora da fare. Forza Italia, che ho oggi l'onore di rappresentare, chiede, d'intesa con le organizzazioni internazionali, di attuare un piano per realizzare in tempi rapidi la riforma del sistema giustizia afghano e i programmi relativi alle infrastrutture e la promozione della formazione. II mio Gruppo, quindi, voterà con convinzione a favore degli ordini del giorno presentati dai senatori Pianetta, Antonione, Mantica e dalla sottoscritta, e alle mozioni dei colleghi della Lega,

colleghe e colleghi, la mozione a firma del senatore Salvi e di altri Capigruppo della maggioranza, che il Gruppo dell'Ulivo si appresta a votare e chiede al Senato di votare, è di grande importanza, a pochi giorni dalla Conferenza internazionale sul sistema giudiziario afghano, che si terrà a Roma il 2 e il 3 luglio prossimi. Un primo merito di questa mozione è di riportare all'attenzione del Parlamento e del Paese un aspetto importante - fondamentale, a mio modo di vedere - della presenza italiana in Afghanistan, che non è solo quella militare, che giustamente sta sempre al centro della nostra attenzione e delle nostre preoccupazioni. È importante riportare al centro dei nostri lavori l'impegno che da cinque anni l'Italia assume in Afghanistan per sostenere la creazione di un sistema di giustizia. Spero che tutti concordino sul fatto che senza giustizia, senza la certezza del diritto, non può esistere la democrazia e innanzitutto il rispetto dei diritti umani. Questa mozione rileva giustamente il ruolo importante, fondamentale e decisivo che l'Italia svolge per il futuro dell'Afghanistan. È altrettanto importante che metta in evidenza l'impegno dell'Italia nel mondo tramite le sue ONG, a dimostrazione della cultura umanitaria e del rispetto dei diritti umani fondamentali che sta nel DNA del popolo italiano. straordinaria degli italiani nel mondo è qui riconosciuta e valorizzata grazie all'impegno di Emergency. È giusto ed è necessario che nel quadro della Conferenza internazionale sul sistema giudiziario afghano si richiami tutti, la comunità internazionale e le autorità afgane, all'applicazione concreta dei princìpi e dei valori che si sono definiti e si continuano a costruire sul piano legislativo. L'impegno italiano e internazionale deve riscontrare da subito effetti positivi e virtuosi sul piano dei diritti umani. alla liberazione di Rahmatullah Hanefi, per il quale il Governo italiano si è giustamente e fortemente impegnato. Va altresì richiamata l'attenzione del Governo afghano sulla drammatica situazione nel penitenziario di Pol-i-Chark. È urgente intervenire, in particolare sulle condizioni di 70 giovani donne e 50 bimbi; ogni giorno che scorre in discussione è un giorno di sofferenza per queste donne e bambini. la nostra solidarietà verso la deputata Malalai Joya è totale, e ci aspettiamo effetti concreti per garantire la sua incolumità e i suoi diritti. È poi doveroso esprimere tutta la nostra preoccupazione per le vittime civili causate dai combattimenti in corso. Questa mozione riconosce l'impegno positivo del Governo italiano, ma anche dell'Italia tutta tramite le sue ONG umanitarie, e sollecita il Governo e tutti noi a intensificare le azioni per aiutare e accelerare, se possibile, il processo di realizzazione e organizzazione del sistema giudiziario in Afghanistan, nel rispetto dei diritti umani. Colleghe e colleghi, nel leggere le varie mozioni presentate mi è tornato in mente un fatto, che in apparenza può apparire non pertinente con l'argomento in discussione, avervi riflettuto, mi sembra molto pertinente; ve lo ricordo brevemente. Nel 2001, in una Conferenza a Berna, ho vissuto un momento che per me si è rivelato una grande lezione di vita. Questa lezione mi è stata data da un uomo che purtroppo ci ha lasciato troppo presto. Molti di voi lo hanno conosciuto: era l'amico Renzo Imbeni, in quel momento vice presidente del Parlamento europeo. In quella veste incontrò a Berna il rappresentante di 600.000 immigrati non comunitari che avevano con l'Europa il problema dei visti di Schengen. L'amico Imbeni fu sottoposto ad un attacco continuo in quella Conferenza, con una domanda che tornava in continuazione: cos'è l'Europa? Cos'è questa Europa che si chiude con Schengen? Questa fu la risposta del Vice presidente del Parlamento europeo: non so cos'è l'Europa, ma so cosa l'Europa non è e non sarà mai. L'Europa non sarà mai uno spazio dove i genitori pensano di essere proprietari dei figli, uno spazio dove l'uomo pensa di essere proprietario della donna, uno spazio dove lo Stato pensa di essere proprietario dei cittadini. Questo l'Europa non lo sarà mai. Bene, colleghe e colleghi, è forti di questi valori che dobbiamo impegnarci per esigere il rispetto dei diritti umani, forti sì di questi valori, ma anche con l'umiltà con l'umiltà di rispettare i valori altrui, e soprattutto con la consapevolezza che noi parliamo di queste tragiche realtà, estremamente delicate e complesse, dalla nostra situazione di comoda sicurezza. Colleghe e colleghi, forti di questi valori, credo che tutti noi dobbiamo fare un passo indietro per far fare un passo avanti all'Italia, per affrontare finalmente la politica estera dell'Italia spoglia da ogni strumentalizzazione

Di questo si tratta e di questo correttamente si deve parlare, come le mozioni stesse ci invitano a fare.

costante, quotidiano, di cooperazione internazionale, affinché l'affermazione dei princìpi fondamentali

la Convenzione contro la tortura, la Convenzione sull'eliminazione di tutte le forme di discriminazione contro le donne, la Convenzione per i diritti del fanciullo, il Patto internazionale sui diritti civili e politici e quello sui diritti economici, la Convenzione sull'eliminazione di tutte le forme di discriminazione razziale, i Protocolli opzionali sui diritti dei fanciulli. L'Afghanistan ha anche ratificato lo Statuto di Roma della Corte penale internazionale il Consiglio dei diritti umani, nel corso della seconda sessione dell'ottobre 2006, ha accolto con soddisfazione la cooperazione del Governo afghano con l'Alto commissariato delle Nazioni Unite

ricordo rapporti di organismi internazionali e di ONG, come Amnesty International, di pochissimi anni fa, che contestavano anche all'Italia la violazione di diritti fondamentali dell'essere umano ed è di pochi decenni fa l'eliminazione nel nostro Paese della scriminante per il delitto d'onore.

Dobbiamo andare orgogliosi di questa attività, compiuta, ad esempio, nei Paesi latinoamericani, dopo le dittature, per la realizzazione anche in quei Paesi di alcuni fondamentali strumenti per l'esercizio della giurisdizione. Questo è, quindi, un lavoro che va compiuto e che continuiamo a svolgere, fermo restando che, in occasione della Conferenza di Roma, l'impegno quotidiano deve essere volto - e va in questa direzione la massima determinazione

Tutte le mozioni hanno sottolineato questi elementi: l'affermazione di alcuni passi in avanti e la necessità di dare concretezza agli strumenti che ho richiamato. Questo è scritto in tutte le mozioni:

in altri termini, sviluppo e sicurezza per il popolo afgano non possono essere raggiunti senza che questo intraveda ragionevoli prospettive di consolidamento della *Governance*, in particolare riferita al settore della giustizia; così, nell'ordine del giorno G1, presentato dai colleghi Pianetta, Antonione e Mantica, vi è l'indicazione della necessità di sforzi ulteriori (si evidenzia, in questo caso nel dispositivo, l'impegno a «superare l'attuale ritardo della riforma del sistema giudiziario afghano, per realizzare l'implementazione delle relative infrastrutture e

nella parte dispositiva credo vi sia un refuso, laddove si parla «del rafforzamento dell'architettura e dei meccanismi internazionali».

Nel secondo capoverso della parte dispositiva, inviterei il collega Salvi ad apportare una modifica al testo, perché il tema della «commissione per la verità e la giustizia»

una situazione di crisi e procedere ad una conciliazione nazionale. La modifica che propongo è pertanto la seguente: «ad adoperarsi nelle sedi internazionali competenti per l'attivazione di ogni utile strumento volto ad affermare verità e giustizia sulla violazione dei diritti umani

di un negoziato politico, una decisione di un tribunale nazionale, dell'assemblea delle Nazioni Unite o del Consiglio di Sicurezza. Mancano elementi di oggettività, e inoltre, voglio ricordare che, ad esempio, un Paese del bacino del Mediterraneo che era considerato in cima alla lista dei Paesi che favorivano il terrorismo, ha sviluppato un'azione che lo ha portato a collocarsi nuovamente nel contesto internazionale anche attraverso un'attività

nella parte delle motivazioni, su illazioni o articoli ripresi da notizie e fonti giornalistiche. C'è l'autorità giudiziaria che sta seguendo

«e adottando ogni necessaria misura al fine prioritario di salvaguardare l'incolumità degli ostaggi». Questo è quanto ha sempre guidato il Governo italiano nelle situazioni che si sono verificate in passato in questi casi. Ancora, nel secondo ed ultimo capoverso,

del Governo, in particolare l'approvazione della linea politica tenuta dall'Italia. Tuttavia, vorrei sottolineare che, almeno a mio giudizio, c'è un punto c'è un punto di merito su cui occorre riflettere, dove nel testo si dice: «dopo cinque anni di impegno della Comunità internazionale in Afghanistan e dopo il conseguimento di importanti risultati (...), la ricostruzione del Paese pare giunta ad una nuova fase». Poiché il significato di questa frase lascia intendere una prospettiva in atto e immediatamente positiva,

Voglio ricordare che questo inciso è il manifesto pubblicato dal Ministro degli affari esteri sul sito della Conferenza proprio a pubblicità dell'iniziativa. *(Applausi

Presidente, non sfugge certo all'acume del presidente Calderoli che sappiamo benissimo di cosa si tratta, conosciamo i problemi.

per costruire una posizione più avanzata del Governo italiano da parte del Parlamento nella Conferenza internazionale; è esattamente questo, collega Calderoli, altrimenti non si comprenderebbe lo spirito di questa discussione. Mi pare ci sia uno scambio di apprezzamenti da parte del senatore Calderoli verso la politica del Governo e da parte del Governo verso la proposta del senatore Calderoli; non vedo dove sia il problema.

in altre sedi e che meriterebbe una discussione approfondita ed organica, in un modo un po' surrettizio. Ho espresso parere favorevole sull'ordine del giorno

quegli emendamenti che potrebbero congruamente essere espressione del dispositivo delle mozioni

disegno di legge n. 1485 si svolge immediatamente dopo la discussione ed il voto sulle mozioni relative agli studi di settore, questione posta all'attenzione del Senato per iniziativa delle opposizioni. Questo è bene sottolinearlo,

fine. Si tratta di tradurre quegli impegni in norme. Tali questioni sono state definite anche con una serie di emendamenti, alcune altre invece rimangono,

C'è poi una questione importante come quella del cuneo fiscale relativo a banche e ad assicurazioni, in cui il Governo fa il gioco delle tre carte e con una mano dà e con l'altra riprende, naturalmente a carico delle stesse banche e assicurazioni, e soprattutto con un'ulteriore violazione delle norme relative allo Statuto del contribuente. Abbiamo ascoltato stamane il Garante del contribuente, che ci ha portato un quadro drammatico della situazione del rispetto delle norme fiscali; signor Presidente, credo che un breve riesame in Commissione del provvedimento potrebbe consentire di ridefinirlo meglio, perché questo è un provvedimento correttivo, ma nella precarietà; noi, invece, vorremmo dare qualche certezza in più rispetto ad una serie di obbligazioni e adempimenti fiscali che rimangono, allo stato, sulla carta,

dare un'ulteriore possibilità al Governo che non è stata esitata - per quanto richiesta, secondo l'opposizione, in maniera compiuta - e cioè di fornire un chiarimento del perché nell'articolo 2 originario del provvedimento si proroghi ancora la possibilità di richiesta di rimborso dell'IVA pagata sulle automobili così come da sentenza della Corte di giustizia europea. Ricordiamo che la sentenza della Corte di giustizia europea ha fatto sì che fosse rivisto in aumento l'indebitamento e quindi il *deficit* dell'anno precedente, portandolo al 4,5 e che invece si rende necessaria, secondo la dichiarazione del Governo, resa dal sottosegretario Grandi, di prorogare ancora la richiesta di rimborso dell'IVA dal 20 aprile a settembre. La giustificazione addotta è che nel momento in cui era stata fatta la proposta di proroga erano state presentate soltanto poco più di 5.000 richieste. Riteniamo che questo sia dovuto al fatto che, essendo stato portato l'acquisto nel passato ad portato l'acquisto nel passato ad ammortamento, la differenza tra quanto è ammortizzato per il bene e quello che potrebbe essere rimborsato dall'amministrazione per i ristori di IVA, dà una lieve differenza per soggetto contribuente da non rendere appetibile appetibile la richiesta. Nel frattempo, però, è accaduto che con posizionamento sotto la linea, come si dice, è stato previsto in tabella B un fabbisogno per regolazione debitoria nel triennio successivo per

quindi si ha una lettura del debito influenzata da una previsione di spesa, di erogazione di cassa che non sta avvenendo e che si sta prorogando nel tempo. Ma perché lo Stato proroga nel tempo la possibilità di richiedere questo ristoro, se il contribuente non ha deciso di farlo? Questo non è chiaro, non è stato chiarito dal Governo entro il in cui il provvedimento è stato all'esame della Commissione, il ritorno in Commissione probabilmente potrà dare questa possibilità al Governo, atteso che si tratta di un provvedimento che, per quanto influenza il mantenimento il mantenimento del debito, ha una grande importanza, anche perché consentirebbe di tracciare meglio il tendenziale, dato che il tendenziale è stato scritto con un 4,5 che a questo punto non è riprovato dalle

che contiene delle normative importanti, tutte a vantaggio, giustamente, del contribuente e molto attese nella generalità delle situazioni, che sarebbe assolutamente controproducente ritardare. Apprezzo molto l'ultima considerazione del senatore Girfatti,

la mozione che abbiamo approvato alcuni giorni fa sugli studi di settore, anche noi siamo molto interessati a che quella mozione abbia effetto ed efficacia, ma questo lo si può fare perché già sono stati presentati emendamenti al testo che possono interpretare quella mozione nella discussione di merito. Soprattutto, grazie all'iniziativa del presidente Benvenuto in qualità di relatore, di concerto con il Governo, e sentiti i colleghi, è possibile che nella discussione si introducano ulteriori affinamenti.

di quel mondo economico per il rilancio dell'economia e dello sviluppo che tutti vogliamo perseguire come obiettivo e come risultato.

concordo con quanto poc'anzi illustrato dal senatore Barbolini: questo provvedimento è atteso dal mondo dell'imprenditoria; parliamo della correzione del grave errore commesso con la norma sugli ammortamenti e poi con il finanziamento dell'IVA sugli autoveicoli, quindi dei problemi della detraibilità. Questo disegno di legge va nella direzione di correggere appunto errori gravi, che hanno anche causato notevoli perdite, soprattutto per quanto riguarda gli ammortamenti nel settore immobiliare. È quindi la dimostrazione dell'improvvisazione della politica fiscale del Governo e di questa maggioranza. Siamo d'accordo sugli articoli del disegno di legge che riguardano gli ammortamenti e l'IVA, ma in Commissione e in Aula presenteremo degli emendamenti che vanno nella direzione ulteriore di correggere - permettetemi il termine - le amenità

abbiamo proposto alcuni emendamenti sulla tracciabilità dei pagamenti e sulla rivisitazione degli studi di settore che vanno proprio nella direzione di quanto è auspicato da parte delle categorie produttive del nostro Paese. Quindi, senatore Barbolini (ma mi rivolgo naturalmente alla Presidenza), è giusto e bello dire che questo provvedimento è atteso dal mondo produttivo, ma sarebbero state attese anche altre iniziative. A questo punto, la giustificazione «ne facciamo pochini» a mio avviso è assolutamente insufficiente:

ulteriore errore della politica fiscale del Governo presa in contropiede. Le proposte Visco di escludere assicurazioni e banche hanno visto l'opposizione giusta dell'Unione Europea

degli sgravi, come è stato notato nella stampa di settore, per le imposte dirette e l'ICI agli edifici rurali delle cooperative.

categorie nuove e specifiche per definire rurali gli edifici delle cooperative; ebbene, questa identificazione, quindi l'assoggettamento alla categoria estesa degli edifici rurali, comporta delle conseguenze di carattere fiscale,

sostenuto che con questo emendamento introdotto all'interno del disegno di legge è stato esteso il raggio degli sgravi per le imposte dirette e per l'ICI. Quindi, signor Presidente, la giustificazione di un provvedimento di correzione che provoca e consente degli aggiustamenti in ordine alla politica fiscale del Governo è insufficiente.

Riteniamo che la risposta sia assolutamente insufficiente e che affermare comunque che una parte di questo disegno di legge va a soddisfare le esigenze del mondo imprenditoriale non sia sufficiente. sia sufficiente. Riteniamo anche che alcuni emendamenti presentati dalla maggioranza e accolti in Commissione abbiano bisogno di considerazioni molto più approfondite in merito alle conseguenze che possono produrre nel mondo delle autonomie locali in ordine all'introduzione nella categoria dei fabbricati rurali di fabbricati di edifici che fino a quando non sarà approvata questa legge non saranno ivi compresi. Signor Presidente, la critica

Presidente, colleghi, l'esame del disegno di legge n. 1485 giunge in un frangente davvero particolare del confronto politico tra maggioranza e opposizione sui temi della fiscalità, nel rapporto tra le politiche antievasive e antielusive e i soggetti contribuenti, cittadini e imprese. Solo poche ore fa - lo si ricordava anche prima - abbiamo concluso un dibattito particolarmente impegnativo sul tema degli studi di settore, un argomento questo, badate, trattato dalla Commissione finanze proprio in sede di esame del presente disegno di legge, con l'approvazione di un ordine del giorno da parte delle forze dell'Unione che poi ha dato origine alla mozione di maggioranza accolta dall'Aula. A mio parere, con il voto di martedì sera si è marcato un cambio di passo per l'azione di Governo, l'azione di Governo, fortemente voluto dalle forze parlamentari di maggioranza, che non intende mettere in discussione il primario obiettivo di una giusta e serrata iniziativa volta a contrastare e combattere l'evasione e l'elusione fiscale. Direi, piuttosto, che si è resa ancora più evidente la consapevolezza che, per meglio affrontare questa sfida, per rendere più equo e moderno il nostro sistema Paese, per recuperare base imponibile e quindi risorse da destinare allo sviluppo e alla stessa diminuzione della pressione fiscale, è necessario operare sapendo promuovere e praticare una fattiva collaborazione, un impegno comune - come si è detto tra lo Stato e la platea dei contribuenti leali, a cominciare appunto dal nostro diffuso sistema di piccole e piccolissime imprese interessate dagli studi di settore. In questo quadro, l'originario disegno di legge n. 1485, volto a introdurre particolari disposizioni attese dai contribuenti in materia di ammortamento dei fabbricati e di rimborsi IVA per le auto aziendali, è stato arricchito dal confronto e dall'esame in 6a Commissione con l'inserimento di modifiche a particolari disposizioni tributarie. Si tratta, infatti, di significativi emendamenti aggiuntivi apportati al testo originario, che mirano a raccogliere la domanda di semplificazione e facilitazione nei rapporti tra il contribuente (famiglie e imprese) ed il fisco. Su questa linea, infatti, si muovono le disposizioni approvate in Commissione finanze e ora all'attenzione dell'Aula. Penso, in particolare, alle modifiche apportate in materia di aggiornamento del catasto dei terreni disposto per il 2007 dal decreto-legge n. sono di particolare importanza, sono molto attese dagli operatori agricoli e tengono conto delle difficoltà emerse. È noto infatti che, una volta notificate le nuove rendite da parte della competente Agenzia del territorio, si sono evidenziate difformità evidenti tra le colture dichiarate dagli operatori agricoli e quelle a loro attribuite dalla procedura informatizzata. Le disposizioni in questione, come approvate in Commissione, consentono quindi ai soggetti interessati di regolarizzare i pagamenti effettuati, con riferimento alle nuove rendite catastali, entro il termine del 30 novembre 2007 e ciò senza applicazione di sanzioni. Allo stesso tempo, è opportuno segnalare che viene differito al 30 settembre il termine per proporre eventuale ricorso. Il disegno di legge in esame, nel testo modificato dalla Commissione, propone inoltre una revisione della disciplina dei fabbricati rurali. Anche in questo caso, si tratta di disposizioni particolarmente significative, attese dalla platea dei contribuenti interessati. Le modifiche legislative proposte sono volte a precisare, ai fini fiscali, le caratteristiche e l'ampliamento degli ambiti di strumentalità di detti fabbricati. Oltre alle predette modifiche, che ho inteso richiamare per la loro indubbia e particolare importanza, ritengo di dovere evidenziare in termini positivi il fatto che la Commissione ha provveduto all'approvazione di alcuni ordini del giorno, accolti dal Governo, finalizzati anch'essi all'individuazione di possibili soluzioni a determinate situazioni, e ciò sempre nell'ottica di dare riscontro all'esigenza di un più positivo rapporto tra Stato e cittadino contribuente. In particolare, segnalo all'attenzione del nostro confronto il testo di un ordine del giorno che impegna il Governo ad un consistente adeguamento della quota deducibile per i figli a carico (ferma dal 1995), da introdurre nella prossima finanziaria con un meccanismo di adeguamento automatico. Esprimo infine un mio personale giudizio positivo su ulteriori emendamenti al testo che il relatore ha presentato all'attenzione dell'Aula. Mi riferisco in particolare agli emendamenti concernenti l'individuazione di nuovi limiti di deducibilità per le auto aziendali dal 2007 e la riduzione del cuneo fiscale per le aziende del credito e dell'assicurazione. Sul primo argomento, va messo in evidenza che, con l'emendamento proposto, si giunge ad ampliare, dopo le limitazioni introdotte dal decreto-legge n. 262 del 2006, la deducibilità dei costi di acquisto e di manutenzione dei veicoli utilizzati da imprese e professionisti non esclusivamente nell'ottica di imprese di lavoro autonomo. Si affronta così un tema particolarmente sentito dalle categorie interessate, che fa seguito all'autorizzazione del Consiglio dell'Unione Europea di consentire la detraibilità al 40 per cento dell'IVA relativa proprio ad acquisti e manutenzione degli stessi veicoli. Sul secondo tema che ho ricordato, l'emendamento proposto dal relatore rappresenta un indubbio passo in avanti rispetto al quadro d'azione definito dalla maggioranza sulla riduzione del cuneo fiscale con la finanziaria per Un passo avanti di sicura importanza, poiché con questa proposta emendativa si provvede a ridurre il cuneo fiscale anche per banche e assicurazioni, superando così le stesse obiezioni sorte in materia in sede europea e dando completa attuazione alla manovra, fortemente voluta da questa maggioranza, tesa a ridurre il peso del costo del lavoro per favorire e rafforzare la competitività del nostro sistema produttivo. Signor Presidente, per il complesso delle disposizioni contenute nel provvedimento e per gli ulteriori elementi modificativi proposti, mi pare quindi che sussistano tutte le motivazioni perché vi sia un positivo accoglimento da parte dell'Aula del presente disegno di legge.

il disegno di legge in esame, sia nel testo originario, sia in quello derivante dalle integrazioni apportate dalla Commissione, introduce una serie di disposizioni fiscali favorevoli ai contribuenti. il piacere di rimarcare come, nonostante le differenziazioni, un obiettivo condiviso ed un positivo clima in Commissione ci abbiano permesso di rafforzare ulteriormente un testo

che, modificando il decreto Bersani-Visco, prevede l'imputazione dellequote di ammortamento già dedotte in misura proporzionale al costo dell'area di costruzione e a quello del fabbricato, consentendo ai contribuenti di utilizzare, per periodi d'imposta successivi, quote di ammortamento dedotte riferibili ai terreni. Ripercorrendo rapidamente il risultato di questo lavoro, vorrei anche sottolineare che l'articolo 3 autorizza la spesa di 5,7 miliardi di euro per ciascuno degli anni 2007, 2008 e 2009, al fine di consentire la liquidazione dei rimborsi delle somme indebitamente versate a titolo di IVA per i veicoli ad uso promiscuo. Di identico carattere integrativo e correttivo sono le norme aggiuntive approvate in Commissione, in particolare quelle dirette a migliorare disposizioni della legge finanziaria 2007, che hanno rivelato, in questi primi mesi di applicazione, profili di criticità, passibili di miglioramento: anche in questo caso, abbiamo costruito norme particolarmente attente alle esigenze dei contribuenti. L'articolo 2 - com'è stato precedentemente ricordato - dà soluzione ai delicati problemi determinati dall'aggiornamento del catasto agricolo. registriamo come l'equilibrata soluzione prospettata dal provvedimento abbia riscontrato una significativa adesione delle associazioni rappresentative degli imprenditori agricoli. La problematica relativa alla revisione dei redditi fondiari è stata oggetto di un ordine del giorno approvato in Commissione, con il quale si impegna il Governo, in caso di disallineamenti dei valori delle rendite fondiarie, a dare disposizione ai competenti uffici dell'Amministrazione tributaria, affinché le istanze in autotutela siano esaminate in via prioritaria, in modo da consentire ai contribuenti, nell'eventualità di una conferma delle effettive rendite catastali attribuite dall'Agenzia del territorio, la puntuale presentazione della dichiarazione integrativa. Viene risolta, inoltre, la questione relativa alla determinazione del tasso convenzionato di cambio, ai fini della tassazione dei redditi dei soggetti residenti nel Comune di Campione d'Italia, correggendo una discrasia emersa tra due norme del decreto Bersani-Visco. L'articolo 5 introduce nuovamente il compenso per i soggetti che prestano assistenza fiscale, anche nel caso in cui il contribuente non sia obbligato alla presentazione del modello unico. Viene inoltre introdotto un elemento di semplificazione escludendo la compensazione di crediti e debiti inferiori a 12 euro. Ripercorrendo velocemente l'articolato, mi soffermerei anche sull'articolo 6, introdotto dalla Commissione, relativo all'esenzione contributiva per alcune categorie di lavoratori dello spettacolo. Prevedere con maggiore chiarezza che giovani, studenti, pensionati e lavoratori, che già versano i contributi, godano fino a 5.000 euro di reddito dalle attività di spettacolo è un piccolo, ma significativo contributo all'autoproduzione culturale e alle figure emergenti dello spettacolo. In tema di fabbricati rurali (è stato ricordato, ma lo ribadiamo), con l'articolo 7 viene consentita l'utilizzazione da parte del soggetto titolare del diritto di proprietà o di altro diritto reale per esigenze connesse all'attività agricola e e viene ampliato il carattere di ruralità alle costruzioni necessarie allo svolgimento delle attività agricole (quali la protezione delle piante, la conservazione dei prodotti agricoli, la custodia di macchine agricole, l'allevamento e il ricovero degli animali, l'agriturismo, l'abitazione dei dipendenti, l'ufficio dell'azienda agricola, la trasformazione ed il maso chiuso). In un contesto di norme attento alle esigenze dei contribuenti, è utile sottolineare, infine, anche l'attenzione all'efficacia e alla buona amministrazione. La Commissione, infatti, ha introdotto una norma volta a modificare l'orario di apertura al pubblico delle conservatorie dei registri immobiliari con conseguente risparmio per il bilancio dello Stato. Chiudo considerando che questo provvedimento semplifica e agevola il rapporto tra contribuente e Stato, ma altra strada dovremo fare su questo terreno. I numerosi ordini del giorno approvati in Commissione indicano un percorso a favore del contribuente a cui siamo sicuri il Governo e la maggioranza, con il concorso dell'opposizione, sapranno dare continuità. Elevare, a partire dalla prossima legge finanziaria, la soglia di reddito al di sotto della quale i familiari sono considerati a carico, introdurre, nell'opera di revisione della disciplina delle tasse dei diritti marittimi, specifiche misure dirette a favorire la maggiore competitività del sistema portuale italiano, reintrodurre l'esenzione IVA per le locazioni di fabbricati ad uso abitativo effettuate in attuazione dei piani di edilizia residenziale convenzionata, dalle imprese costruttrici o dalle imprese che hanno effettuato interventi di recupero edilizio ed eliminare l'aliquota IVA, intervenire in materia di agevolazioni fiscali sugli impianti di teleriscaldamento, semplificare la disciplina relativa all'obbligo di presentazione dell'elenco dei clienti e dei fornitori, sono solo alcuni degli interventi che la Commissione ha indicato come interventi che da subito possono essere realizzati.

di intervenire non si sia adottato lo strumento più idoneo, che è quello del decreto-legge. La maggioranza, Presidente, ha presentato ben dieci ordini del giorno che costituiscono altrettante richieste di intervento legislativo. Il consenso registrato in Commissione rispetto all'intervento modificativo e correttivo del decreto-legge n. 223 del 2006, prevedendo l'imputazione delle quote di ammortamento già dedotte in misura proporzionale al costo dell'area di costruzione e a quello del fabbricato strumentale, non deve nascondere le questioni di politica tributaria che emergono in tutta la loro gravità. Non avevamo mancato di sottolineare la rozzezza di alcune scelte operate, peraltro con effetto retroattivo, dai decreti Bersani-Visco, che hanno determinato effetti negativi nel sistema economico e penalizzanti per altri settori, per esempio per il ricorso al *leasing* quale strumento principale per gli investimenti in tale settore. E come non porre attenzione rispetto alla vicenda delle SIIQ e alle relative preoccupazioni già espresse in legge finanziaria per i rischi che stanno emergendo rispetto alla traslazione delle minusvalenze, onorevole Sottosegretario, sui risparmiatori, con i conflitti di interesse tra SGR e SIIQ, cioè società di investimento immobiliare quotate. Il provvedimento prevede l'appostazione della copertura finanziaria per i rimborsi delle somme indebitamente versate a titolo di imposta sul valore aggiunto per i veicoli ad uso promiscuo, anche se si registrano forti ritardi nell'applicazione della norma e quasi un tentativo di «stancare» i contribuenti che stanno preferendo la strada dell'abbandono piuttosto che un percorso tortuoso e costoso. Con un emendamento, credo dell'ultima ora, si corregge ulteriormente tale normativa, però intervenendo con ulteriori limiti. Non si può non sottolineare il quadro di incertezza e di forti perplessità rispetto al calendario delle scadenze tributarie con un provvedimento del direttore dell'Agenzia delle entrate. Ormai, signor Presidente, siamo alla "comunicazione legislativa" da parte dell'Agenzia. Ribadisco la priorità dell'obiettivo di assicurare la certezza del diritto e la irretroattività delle disposizioni tributarie nella elaborazione della normativa fiscale e convengo sulla esigenza, da molti prospettata, di una celere approvazione di questo provvedimento, che non può però essere disgiunta da un esame più compiuto, più attento, più sereno, più produttivo. Ho presentato una serie di proposte emendative, tra le quali una in tema di revisione delle rendite catastali dei terreni agricoli; una soluzione più adeguata rispetto all'incertezza determinata dalla soluzione della maggioranza, che produce solo precarietà. L'aggiornamento della qualità di coltura catastale è infatti avvenuto sulla base delle affermazioni contenute nelle domande di accesso ai contributi agricoli comunitari, con procedure automatiche. Si è pertanto proceduto all'adozione di specifiche tabelle di corrispondenza tra le circa 700 specie vegetali (colture dichiarate nelle domande di finanziamento) e le circa 100 qualità di coltura catastale di riferimento. L'adozione di meccanismi automatici nella variazione delle colture iscritte negli archivi catastali ha determinato una serie di difformità tra le colture effettivamente praticate e quelle iscritte nel catasto. Pertanto la procedura di revisione, fondata sull'indiscriminato incremento delle rendite catastali, ha determinato effetti penalizzanti per i redditi agricoli dominicali correlati con il pagamento delle imposte immobiliari. Tutto ciò resta nell'assoluta incertezza rispetto alla scadenza tributaria, perché stiamo esaminando un disegno di legge in un mese di scadenze tributarie. Un ulteriore profilo di criticità è rappresentato dalle modalità con le quali l'Agenzia del territorio ha pubblicato l'elenco dei Comuni per i quali era stata attuata la rivalutazione dei redditi agricoli. dei redditi agricoli. Al riguardo, in luogo della pubblicazione sulla *Gazzetta Ufficiale*, avvenuta in deroga alla normativa vigente, sarebbe stata più corretta una forma di notificazione personale, anche al fine di consentire agli interessati la possibilità di valutare tempestivamente l'eventuale presentazione di un ricorso. Su tale specifico profilo c'è la sovrapposizione della scadenza (al 1° giugno 2007) del termine per presentare ricorso con il periodo di tempo previsto per la denuncia dei redditi e dell'ICI direttamente correlata alle revisioni effettuate. Durante lo svolgimento di uno specifico atto di sindacato ispettivo presso l'altro ramo del Parlamento, l'Agenzia del territorio ha confermato la sussistenza di situazioni di difformità tra il dato catastale e quello reale, riconducibili al fatto che il procedimento di rivalutazione delle rendite è stato condotto sulla base di criteri teorici, se non addirittura virtuali. Atteso l'apporto fornito sul piano tecnologico dalla SOGEI alla realizzazione dell'intervento, considerando anche la collaborazione prestata da tale società quale indiscutibile valore da preservare per il miglioramento della efficienza dell'amministrazione tributaria, gli ambiti di attività della stessa SOGEI richiedono una definizione più puntuale degli indirizzi amministrativi da parte delle autorità tecniche del settore. D'altro canto, va negativamente rimarcato anche il fatto che la revisione delle rendite colturali ha effetto a partire dall'anno di imposta del introducendo quindi l'ennesima disposizione tributaria di carattere retroattivo. Altro che Statuto del contribuente! Questa mattina abbiamo ascoltato il Garante del contribuente

dell'*Authority*, in questo senso, perché viene subordinato all'organo che dovrebbe controllare. Rispetto alla complessa problematica appena illustrata, l'emendamento che ho presentato propone una proroga della decorrenza della rivalutazione dei redditi catastali per consentire agli imprenditori agricoli interessati la possibilità di valutare le opportune iniziative anche in sede di autotutela, che - come è stato evidenziato stamattina - non viene esercitata attraverso un maggiore dialogo tra le agenzie, per esempio, tra l'Agenzia del territorio e l'Agenzia delle entrate, ma ognuno va per proprio conto e il cittadino contribuente viene abbandonato a se stesso. Un'altra questione che merita di essere affrontata in questa sede è l'accesso ai passi carrabili nei fondi rustici. Affrontiamo un problema e non viene affrontato in modo adeguato per le problematiche che sono insorte dopo l'apertura di un contenzioso tra tra ANAS ed enti locali, in particolare con le Regioni Puglia e Piemonte. Il problema della sicurezza degli accessi nelle strade, soprattutto nelle aree interne, non può essere scaricato sulle imprese agricole in particolare quando ci sono più accessi come avviene nelle aree di montagna e nelle aree interne. Altre modifiche riguardano la disciplina dell'ammortamento dei fabbricati adibiti ad immobili strumentali nell'esercizio di una attività produttiva. Emerge l'esigenza di apprestare un rimedio all'impianto sotteso al decreto Bersani-Visco, errato in quanto fondato su un'analisi non corretta del quadro informativo. Tale osservazione rinvia all'erronea impostazione della manovra di finanza pubblica in generale, che determina effetti depressivi per il sistema economico, come dimostrato anche dai dati degli ultimi tre mesi sull'andamento delle entrate tributarie. Le proposte preannunciate sono volte a confermare l'esenzione fiscale per i fabbricati ad uso abitativo o anche destinati ad uso diverso, nonché il mantenimento del regime IVA previsto sulle operazioni immobiliari effettuate entro l'arco di un quinquennio nella prospettiva di incentivare gli investimenti per le ristrutturazioni edilizie. Avete dato risorse alle SIIQ, che ho prima citato, perché lì naturalmente si tratta degli amici degli amici (quella storia la tireremo fuori quando sarà il momento opportuno), ma non fate nulla per la cedolare secca per gli affitti che pure era un impegno elettorale del vice presidente del Consiglio Rutelli. Come non fate nulla per favorire il recupero del patrimonio edilizio di interi immobili, mentre la misura agevolativa per le singole unità immobiliari è stata più volte prorogata nel corso degli anni in favore delle persone fisiche, perfino nell'ultima finanziaria. La detrazione non è stata prevista anche per gli interventi di restauro e di ristrutturazione edilizia eseguiti da imprese di costruzione o da cooperative edilizie. Non fate nulla per estendere il particolare regime agevolativo previsto per l'imposta di registro, le imposte ipotecarie e catastali anche alle cessioni di immobili e piani urbanistici particolareggiati dirette ad attuare programmi di edilizia residenziale, a condizione che sia presente una quota di edilizia convenzionata con le Amministrazioni comunali. Tale proposta rappresenta un idoneo sostegno alle fasce sociali con basso reddito, che non possono procedere all'acquisto di abitazioni ai prezzi di mercato per la bolla immobiliare, ponendo attenzione soprattutto ai giovani, alle giovani coppie, alle aree di più forte disagio, alle aree metropolitane. Assistiamo al paradosso che nei giorni scorsi approvate in Commissione finanze l'atto di l'atto di indirizzo per il conseguimento degli obiettivi di politica fiscale per il triennio 2007-2009 e alcuni rappresentanti della stessa maggioranza scrivono al Presidente del Consiglio per lamentare la scarsa attenzione al problema degli studi di settore.

Ribadisco, inoltre, le osservazioni critiche già formulate sulla circostanza che nell'adozione delle tabelle di corrispondenza siano stati privilegiati criteri eccessivamente astratti, che non tenevano adeguato conto della realtà delle colture praticate, mentre sarebbe stata preferibile una proroga al 2008 delle disposizioni. Registro criticamente, signor Presidente, l'atteggiamento negativo della maggioranza e del Governo sugli emendamenti presentati dalla mia parte politica (ma anche dall'intera opposizione), che miravano a correggere e migliorare le misure fiscali introdotte dal Governo nell'ottica di favorire i nuclei familiari e i ceti socialmente più deboli. In tale direzione andavano infatti le proposte relative alle agevolazioni per l'edilizia residenziale convenzionata, alla reintroduzione della detrazione di imposta del 36 per cento per le ristrutturazioni di interi fabbricati abitativi, alla proroga degli effetti fiscali della revisione del catasto agricolo, ribadendo sul totale punto di vista l'urgenza del problema degli accessi a pagamento dei fondi agricoli sulle strade di competenza dell'ANAS, che deve essere definita in questo provvedimento con un intervento legislativo. Ribadisco le ragioni che militano a favore di un *iter* veloce, dal momento che il disegno di legge in esame introduce norme che correggono errori fatti dal Governo e da questa maggioranza; misure approvate con un eccesso di precipitazione. Il Governo, signor Presidente, è distante dai problemi del Paese. Come si fa a dire, come ha fatto il vice ministro Visco, che l'introduzione del principio del contrasto di interesse è «una balla colossale»? Porteremo all'infinito questa cosa. Un contrasto di interesse che viene praticato negli Stati Uniti d'America, che vengono presi a modello in tutto il mondo come sistema fiscale efficiente, viene definito «una balla colossale». Come si fa a non comprendere che la questione degli studi di settore sta creando grande preoccupazione tra gli operatori economici? Quelle modifiche devono essere introdotte in questo provvedimento se vogliamo dare esecuzione all'atto di indirizzo approvato martedì scorso.

non ha prodotto nulla e quindi voi state producendo illusioni della stessa componente della maggioranza, che stanno insistendo per ulteriori modifiche. Quindi, siamo favorevoli di consentire il pagamento delle imposte con un allungamento dei termini, senza l'applicazione delle maggiorazioni previste per tutti i soggetti ricompresi nell'area di operatività degli studi di settore. Tuttavia, lamento il mancato ricorso, da parte del Governo, a quel metodo doveroso della concertazione nell'opera di revisione di questo strumento. Non vorrei che le categorie venissero ingannate ulteriormente. In tal senso, il Governo sembra avere ripudiato quel criterio che era stato adottato nella precedente legislatura, diretto a privilegiare un maggiore coinvolgimento delle associazioni di categoria nell'elaborazione del sistema di accertamento dei redditi. C'è il rischio, infatti, che questa nuova disciplina possa dar luogo ad un aumento delle attività di verifica per effetto degli indici di coerenza e di normalità economica che avete introdotto e che appaiono eccessivamente oscillanti, tant'è che oltre il 50 per quello che voi avete prodotto. Tutto ciò richiede scelte precise già in questo provvedimento su punti qualificanti, in particolare la irretroattività delle norme fiscali soprattutto per gli studi di settore, una piena aderenza allo Statuto del contribuente, che viene ulteriormente violato in questa norma che riguarda il cuneo fiscale per banche e una rimodulazione delle scadenze fiscali, e quindi delle scadenze degli operatori, la sperimentatività degli stessi indici,

perché finora sono state dette troppe parole e sono stati praticati pochi fatti.

dopo una fase sperimentale di applicazione, per un verso di norme contenute nel decreto Bersani-Visco e nella finanziaria e, per un altro verso

c'è la possibilità, la necessità e l'urgenza di intervenire per coprire tali carenze di organico e che quindi è necessario provvedere. Al di là delle opinioni e dei pareri espressi dalla 5a Commissione permanente, credo che si riconosca da parte dell'Agenzia del demanio e, quindi, evidentemente da parte del Governo, da parte dei giovani che hanno partecipato al concorso e che ne hanno il diritto, la possibilità, oltre che la necessità, di vedere coronata la prova

costruendo eventualmente assieme le soluzioni più adeguate affinché si dia una risposta positiva a coloro che sono in lista di attesa per un contratto di formazione lavoro.

Il primo modifica il calcolo delle quote di ammortamento deducibili degli immobili strumentali previsto dal cosiddetto decreto Bersani-Visco del 2006, in modo che le quote di ammortamento dedotte nei periodi di imposta precedenti, calcolate sul costo complessivo, siano riferite proporzionalmente anche al costo dell'area e non solo al costo del fabbricato. norma risulta favorevole al contribuente, in quanto consente l'utilizzo, per periodi di imposta successivi, delle quote dedotte in ammortamento per la parte riferibile al terreno. Rimane, tuttavia, in essere la disposizione del comma 8 dell'articolo 36 del decreto-legge n. 223 del 2006 che con superbia decisionale deroga alla efficacia temporale della norma tributaria prevista in materia di Statuto dei diritti del contribuente, in base al quale le disposizioni tributarie non possono avere effetti retroattivi per non turbare quel clima trasparente ed egalitario che lo Statuto assegna al contribuente nei suoi rapporti con il fisco. Ma i Governi spesso se ne dimenticano. L'articolo 2 autorizza la copertura finanziaria alla spesa che permette all'Agenzia delle entrate la liquidazione dei rimborsi dell'IVA pagata in più per l'acquisto o per l'importazione di ciclomotori, di motocicli e di autovetture e autoveicoli adibiti ad uso pubblico o che formino oggetto dell'attività propria dell'impresa, ovvero all'acquisto o importazioni dei loro componenti e parti di ricambio. Tale articolo deriva dalla sentenza della Corte di giustizia della Comunità Europea che rileva una mancata procedura di consultazione del Comitato IVA previsto dalla VI direttiva del Consiglio, relativamente alle proroghe del regime di indetraibilità. Pertanto, la sentenza riconosce il diritto di ottenere il rimborso dell'IVA versata e non detratta negli anni successivi al 2000 per un ammontare di 5.700 milioni per ciascuno degli anni 2007, 2008 e 2009. È ovvio che siamo favorevoli ai due articoli, ma delusi per il risultato della 6a Commissione dove il relatore aveva prospettato la possibilità, tramite questo *iter* parlamentare, di realizzare interventi significativi. Infatti, preso atto della portata di carattere integrativo e correttivo dell'intervento attuato con il presente disegno di legge, sussistevano le condizioni per una sua approvazione in termini brevi per salvaguardare le posizioni soggettive dei contribuenti interessati, e invece ci avviciniamo al sessantesimo giorno di giacenza del provvedimento in Senato. In secondo luogo, si chiedeva alla Commissione di valutare l'opportunità di introdurre in modo mirato alcuni emendamenti svolti a correggere la legge finanziaria per il 2007, considerate le criticità emerse in questi primi mesi di applicazione delle disposizioni in essa recate e formulate da ogni settore della vita pubblica, in particolare dal comparto del lavoro nella sua accezione più generale. Sono attese condivise, ma non attuate, sebbene anche l'opposizione si sia adoperata nel proporre emendamenti limitati nel numero per favorire l'intenzione positiva positiva dello stesso relatore, con lo scopo di razionalizzare talune incongruenze normative sussistenti nella legislazione prodotta dall'attuale maggioranza parlamentare. La Commissione, infatti, non ha avuto il coraggio di spingere quest'opera chiarifìcatrice e di armonizzazione del quadro normativo sulle tematiche che la minoranza parlamentare aveva individuato con idonee proposte solutorie aventi lo scopo di evitare un possibile arbitrio interpretativo dell'amministrazione, successivo peraltro ai comportamenti tenuti dal contribuente e per ciò stesso foriero di controversie. Il diniego è stato netto con una ormai abusata richiesta del rappresentante del Governo di trasformare gli emendamenti in ordini del giorno, perpetuando la tiritera del «sì, avete ragione, è giusta la proposta normativa, ma dobbiamo verificare con gli uffici» e, aggiungiamo noi, quando il «potere amministrativo lo permetterà, se lo consentirà, si attueranno le norme contenute in quegli ordini del giorno sicuramente approvati dall'Assemblea». Gli emendamenti che si aggiungono all'articolato originale sono poca cosa e non mitigano la tronfia finanziaria Prodi del 2007 che, con i suoi 1364 commi, rimane l'esempio massimo di un malgoverno normativo di cui nessuno aveva necessità.

perché è opportuno utilizzare questo provvedimento per offrire certezza ai contribuenti, con particolare riguardo alla norma di applicazione dell'inversione della prova nel caso di scostamento degli indicatori di normalità, o, meglio ancora con riferimento alla non retroattività degli stessi indicatori. Per quanto concerne l'articolo 1 sull'ammortamento fabbricati, ci troviamo di fronte ad una norma correttiva dell'ingegneria tributaria, sempre così lontana dalla trasparenza e chiarezza, che fa tornare alla mente il detto di Bastiat che una norma è rispettata se rispettabile: figuriamoci poi quando occorre una norma interpretativa o che rettifichi la precedente. Per quanto invece concerne la disposizione dell'articolo 2 in materia di rimborso IVA sulle auto, è opportuno inquadrare brevemente in quale contesto si pone il provvedimento da cui trae origine l'attuale norma. Con decreto del Presidente della Repubblica n. 633 del 1972 viene introdotta in Italia la istituzione e la disciplina dell'imposta sul valore aggiunto e all'articolo 19-*bis* - siamo nel 1972 - la disposizione sulla indetraibilità di cui ci stiamo occupando. Fu un periodo, quello degli anni '70, caratterizzato dalle difficoltà sorte sulla battuta di arresto della grande espansione postbellica, contraddistinta dalle prime rivendicazioni salariali nei confronti di una dirigenza imprenditoriale che cercava di mantenere il vantaggio dei bassi salari il più a lungo possibile e da una illusione di imitare il sistema fordista americano. Più che imitare si attuò il vezzo di scimmiottare le altrui decisioni in quanto la non collaborazione fattuale fra sindacato ed industriali non portò alla realizzazione americana che aveva ottenuto risultati imbattibili di produttività, correlati a salari più alti, con basso e circoscritto tasso di rivendicazioni salariali. Alle note tensioni del 1969, e ad altro ben noto, seguì la crisi petrolifera che quadruplicò il prezzo del petrolio e conseguentemente aumentarono i prezzi delle materie prime, facendo saltare l'equilibrio faticosamente raggiunto nella nostra bilancia dei pagamenti con un PIL, nel 1975, che toccò un massimo storico di diminuzione del 3,60 per cento per fortuna imbattuto. Erano gli anni dove l'Europa soffriva anche per l'abbandono del regime dei cambi fissi avvenuto fra il 1971 e il 1973 con la dichiarazione della inconvertibilità del dollaro. L'imprenditoria, la piccola e media impresa, reagì e creò quel microrganismo aziendale che con i distretti industriali e l'italica inventiva si insinuò nella internazionalizzazione degli scambi attraverso il *made in Italy*. Anche lo Stato reagì attraverso l'approvazione dello Statuto dei lavoratori e, e, come se fosse solido nei conti, iniziando l'espansione del debito pubblico, con un insieme di provvedimenti sul *welfare state* che diedero corso ad un aumento delle pensioni, alla tutela della disoccupazione, della maternità e così fino alla istituzione del Servizio sanitario nazionale, nato purtroppo obsoleto. Proprio in quegli anni si costruiva il MEC che, fra l'altro, trasferiva nel nostro Paese l'IVA, un'imposta propria delle legislature europee. La legge istitutiva dell'IVA si innestava in un contesto di transizione della nostra pubblica amministrazione che si era formata nel passato regime, ma che anche nello Stato repubblicano continuava ad usare quella metodologia sui registri contabili muniti di sigillo sabaudo e logo del fascio, e applicava la normativa dell'IGE e della Imposta Conguaglio, gestite con ampia tolleranza rispetto alla nuova norma dell'IVA, norma comunitaria che non era stata pensata in Italia né aveva avuto l'apporto di quella burocrazia che doveva applicarla. Ricordiamo che, in quel periodo, una delle norme a vantaggio della nostra economia consentiva la restituzione dei diritti all'esportazione sul valore riferito ai prezzi del listino depositato presso la Camera di commercio. Si aveva, così, un prezzo del mercato interno che spesso era un quinto di quello dichiarato per il rimborso, concedendo all'esportatore di incassare l'equivalente dell'imposta conguaglio all'importazione, cioè il 6 per cento sul valore indicato nei listini. Con l'introduzione dell'IVA questo aiuto alla nostra esportazione veniva soppresso per adeguamento alle norme dell'Europa che, fra l'altro, mal tollerava le incongruenze italiane dovute ad un continuo cambio dei Governi, cambio che a sua volta generava una non adeguata partecipazione della nostra Amministrazione pubblica al diritto comunitario ascendente. Con l'introduzione dell'IVA, inoltre, furono aboliti i dazi comunali i cui dipendenti furono immessi, senza preparazione alcuna, nelle allora Direzioni Generali del Ministero delle finanze, abbassando la qualità professionale dei controlli erariali e generando confusione, di cui si pasce l'evasione. La VI direttiva europea, quella cui si riferisce il nostro provvedimento, fu recepita dall'Italia nel 1979 e all'articolo 17 stabilisce che per motivi congiunturali uno Stato può escludere in tutto o in parte dal regime di deduzione IVA la totalità o parte dei beni di investimento o altri beni. Non solo ancora oggi siamo in perenne congiuntura, ma subiamo sentenze negative sull'operato dello Stato perché la nostra burocrazia non esige dai Governi il rispetto degli accordi, come quello citato, che avrebbe richiesto un comportamento procedurale, a cui, peraltro, sono ricorsi con esito positivo Regno Unito, Austria e Germania. Poiché solo di recente la suddetta procedura è stata richiesta a Bruxelles, l'abbattimento della detraibilità, qualora accordata, consentirà allo Stato di ridurre la perdita del gettito dell'IVA. Ma ricordando la su accennata procedura dei rimborsi all'esportazione sul prezzo di listino delle merci nazionali, siamo convinti che sarebbe opportuno mantenere l'agevolazione sui beni strumentali in quanto è acclarato che meno tasse vengono applicate agli strumenti di lavoro del mondo della produzione e più aumenta il PIL, e con esso più benefici ai cittadini. Abbiamo ricordato a noi stessi alcune fasi del nostro passato in quanto l'analisi di questo provvedimento non può essere limitata al solo comparto fiscale. Riteniamo, infatti, che le misure legislative che gravano sui contribuenti vanno considerate e collocate in un contesto più ampio dove la circolazione dei prodotti e dei fattori deve essere compatibile con la cosiddetta *Way of Life* del mondo occidentale per rendere sostenibile la triade di Dahrendorf: democrazia, coesione sociale e crescita economica. Le notizie che ci vengono dai recenti incontri dell'Unione Europea, purtroppo confermano le nostre preoccupazioni sul ruolo dell'Italia nel consesso internazionale dove Francia, Germania e Regno Unito impongono il loro dettato, mentre noi siamo svelti nel risolvere i nostri problemi economici imponendo tasse su coloro che sono facilmente individuabili. Abbiamo difficoltà ad avere fiducia in chi ci sta vicino, manchiamo di quella speranza nel futuro che lo Stagirita definiva un sogno ad occhi aperti e siamo costretti a rincorrere i nostri *partners* europei con la modestia a cui ci relega questo insipiente Governo. Diamo per scontata la buona fede di chi fa politica ovunque si collochi nell'arco parlamentare,

attua pesanti tagli al sistema dell'istruzione e della ricerca, in particolare dell'università. Devo constatare purtroppo, con grande rammarico, che il relatore né nel suo intervento né nella sua relazione ha fatto alcun cenno ad una resipiscenza, ad una autocritica,

Devo anche aggiungere che il ministro Mussi, in una lettera inviata al presidente Prodi e al ministro Padoa-Schioppa, ha chiamato in causa direttamente il Governo; ha parlato di una responsabilità del Ministro dell'economia di una corresponsabilità dell'intero Governo e del Presidente del Consiglio. Allora è evidente che si apre anche un caso politico: qui denuncio un palese contrasto, un caso politico che deve essere in qualche modo risolto e posto all'attenzione dell'Assemblea. Devo anche aggiungere che il fatto è molto più grave di quanto evidentemente il Governo e la maggioranza non hanno dimostrato di voler considerare, perché - cito soltanto un dato estremamente significativo - in attuazione della finanziaria, l'edilizia universitaria ha già subito un pesantissimo taglio di risorse da 100 milioni di euro a 35 milioni di euro. 35 milioni di euro. Pensate che solo per il 2007 le università si sono già impegnate per ben 80 milioni di euro proprio sul fronte dell'edilizia universitaria. C'è stato un accantonamento di oltre 200 milioni di euro a danno dell'università; con questo taglio al fondo di finanziamento ordinario noi ritorniamo alle somme del 2005.

di una quota estremamente significativa il contributo all'università e alla ricerca. Tra l'altro, il mese di giugno porta evidentemente sfortuna dall'inizio della legislatura all'università italiana, perché nel mese di giugno dello scorso anno venne presentato l'allora decreto Bersani (poi la prima legge Bersani), che tagliava proprio sulle spese intermedie: un taglio di 250 milioni di euro sulle spese di funzionamento delle università, tra l'altro tagliando sulle risorse proprie del sistema universitario. Credo che questo Governo e questa maggioranza dimostrino per un'ennesima volta non solo un disinteresse ma una vera e propria avversione, un odio sistematico manifestato in ogni provvedimento che tocca il sistema dell'università e della ricerca nei confronti di questo delicatissimo e importante comparto. Chiedo allora al ministro Mussi di intervenire per fare, con noi opposizione, una battaglia per cancellare questo emendamento e ribadisco che, nell'ipotesi in cui questa copertura finanziaria non venisse del tutto eliminata, il ministro Mussi dovrebbe a questo punto rassegnare le dimissioni perché un Ministro troppo debole